*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per farle una richiesta e le chiedo di consentirmi di contestualizzarla con cinque concise osservazioni. La richiesta si riferisce all'episodio su cui ha riferito ieri all'Assemblea il collega Paragone, ovvero al fatto che siano stati rimossi

Google non è un monopolista nei servizi in *cloud* ed è abbastanza sorprendente che tenga a far sapere ai suoi clienti che i dati non sono in sicurezza e svegliandosi domattina potrebbero non trovarli. Faccio un rapidissimo inciso personale e me ne scuso. È grazie a Google che io sono grazie a Google che io sono qui, perché Google ha ospitato quel *blog* che, dandomi visibilità nel dibattito, mi ha consentito l'onore di essere vostro collega. È quindi molto strana questa decisione e, da utente soddisfatto di Google, domani cercherò alternative sul mercato. Un altro tema che sottopongo a tutti voi è il seguente: dove vanno a finire i dati quando succede una cosa di questo tipo? Un video contiene anche reazioni e commenti degli utenti, che potrebbero essere conservati ed utilizzati a fini di profilazione politica. Interpellerò in merito l'Autorità garante. Un terzo punto rapidissimo: ricordiamoci che «Eppur si muove», ai suoi tempi, quattro secoli fa, era una *fake news*. Dieci anni fa «l'austerità fa male» era una *fake news*, ma solo su ByoBlu chi voleva argomentarla poteva trovare spazio il Paese dovrebbe essere grato a chi ha consentito di anticipare i tempi del dibattito, dicendo dieci anni prima quello che oggi ci ricorda il signor Presidente del Consiglio dei che sia motivo di orgoglio per tutti noi: dal 24 marzo è finalmente operativa la *web tax*. Questo significa che l'Italia è riuscita a imporre una norma di civiltà ai giganti del *web*, dove l'Europa è ancora in ritardo (OCSE) in grande ritardo. Si può avere perciò a livello di Stati nazionali un'interlocuzione; approfittiamone per una riscossa di civiltà non solo sul piano fiscale, ma anche su quello dei diritti fondamentali, come quello della libertà di espressione. Arrivo alla richiesta, ringraziandola per il tempo che mi ha accordato. Siamo un ramo del Parlamento sensibile a questi temi, guidati da una giurista sensibile e illuminata come lei; le chiedo di poter incardinare un dibattito su di essi che possibilmente giunga a una risoluzione o comunque ad un atto di indirizzo del Governo in questo ambito, favorendo anche l'*iter* di un disegno di legge su questa materia che come contenuto minimo dovrebbe avere, come verificherò con il collega Moles, la richiesta di sottrarre e di schermare le testate giornalistiche registrate che sono sul *web* dal meccanismo delle segnalazioni, che sono il meccanismo utilizzato dalle squadracce digitali degli *hater* organizzati per far rimuovere i contenuti a loro sgraditi. *(Applausi)*. Senatore Bagnai, la ringrazio per aver posto all'attenzione dell'Assemblea un tema così importante, che porrò all'attenzione della prossima Conferenza dei

in un momento difficilissimo e particolare. Stiamo parlando infatti dell'abilitazione all'esercizio della professione forense dei difensori dei diritti dei cittadini, ma prima ancora dei custodi dei diritti dei cittadini, che in questo momento sono compressi e talvolta anche compromessi. Questo è infatti un momento del tutto straordinario, qualcosa che mai avremmo pensato di dover elaborare per questa nobile professione, tra l'altro l'unica costituzionalmente garantita. Per la prima volta dal Dopoguerra, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che già sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021. Purtroppo, a fronte di una diffusione del contagio del virus, che nonostante l'avvio della campagna vaccinale e l'implementazione della stessa non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto, nell'autunno scorso, a disporre il rinvio della prova scritta permangono tuttora. In particolare, le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni sanitarie disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, in particolare nelle sedi metropolitane, di assembramenti, per il numero esorbitante di candidati, per un tempo molto prolungato, quale quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati scritti. In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente nei tre giorni, nelle varie sedi distrettuali del territorio nazionale, in alcuni casi riuniscono migliaia di candidati: penso agli oltre 4.000 nel mio distretto di Corte d'appello, quello di Napoli, ai 3.000 di Milano o ai 3.000 nel distretto di Roma. Ciò non è ragionevolmente possibile, per una serie di considerazioni. L'attuale normativa consente di riunire in un'unica sede non più di 30 persone e dunque o si ricorre a sedi in cui si possano suddividere i candidati in classi di 30 o bisognerebbe trovare soluzioni logistiche, che non sembrano sempre attuabili. L'impegno del personale di controllo sarebbe notevole, in considerazione della pluralità delle sedi. Il rischio connesso al contagio è elevato, così come le difficoltà logistiche e organizzative: pensiamo soltanto alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, alle attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi, considerato che le prove scritte durano sette ore, alla presenza di donne con necessità di cura dei propri figli e di allattamento, a candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio da coronavirus. Tra l'altro, il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento al Comitato tecnico-scientifico, insediato presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo stesso Comitato ha risposto di ritenere che non è possibile, allo stato, lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione per questa sessione, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle prove e delle criticità rappresentate, legate alle difficoltà di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 3 febbraio 2021. Un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a termine poi le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021, Il decreto-legge n. 31 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato in sede referente alla 2a Commissione giustizia, muove quindi dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che rendano possibile, in questo e solo in questo attuale contesto emergenziale, dovuto alle recrudescenze della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense. Ricordiamo che queste prove dovevano già tenersi nel dicembre scorso; un esame che - è opportuno evidenziarlo - secondo le stime del Ministero riguarda circa 26.000 aspiranti avvocato. Per la sessione di esame 2020, ai sensi dell'articolo 1, è stata introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatorie del tutto straordinaria rispetto a quella prevista a regime. L'articolo 2 esclude, per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno, la possibilità di svolgere prove scritte. I candidati sono chiamati quindi a sostenere due prove orali. La prima prova orale sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica e ha ad oggetto la discussione di una questione pratico-applicativa, dove il candidato è chiamato a fornire la soluzione di un caso che richiede padronanza di diritto, sia sostanziale che processuale, in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra materie regolate dal codice civile, materie regolate dal codice penale o diritto amministrativo. Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro della giustizia, previsto nei trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. del decreto-legge. Una seconda parte è dedicata alla discussione orale, conclusa la quale la commissione si ritira in Camera di consiglio per comunicare l'esito della prova al candidato. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prima prova un punteggio di almeno 18 punti. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito. Anche la seconda prova orale è pubblica e deve durare tra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato, svolgendosi almeno trenta giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere circa brevi questioni relative a cinque materie optate preventivamente. Lo stesso candidato deve dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato. Per la valutazione della seconda prova orale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle cinque materie, come per quella avente ad oggetto la deontologia e l'ordinamento. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie. Il testo disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame: per consentire di svolgere le prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni

Il presidente deve essere un avvocato; possono far parte delle commissioni d'esame per la prima volta i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.

Per la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della commissione. Nel caso della seconda prova orale, invece, la modalità di partecipazione della commissione da remoto è facoltativa. L'articolo 5 del testo dispone circa la verbalizzazione della prova d'esame e vi è anche un riconoscimento dei compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni,

abbiamo ritenuto, seppure con un *timing* molto ristretto, di procedere ad un significativo esame, in un'interlocuzione proficua tra tutti i Gruppi parlamentari, seguendo con attenzione ed interloquendo con gli auditi, le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione emergenziale nella quale ormai da più di un anno siamo costretti a vivere ha imposto a tutti noi una rimodulazione della nostra quotidianità, una lotta costante con cui ognuno di noi nel nostro piccolo è costretto a confrontarsi. Molteplici sono stati gli interventi che la politica ha dovuto adottare al fine di fronteggiare e superare questo difficile periodo. Certamente, la sospensione dell'esame di abilitazione

gli enormi sforzi di circa 26.000 aspiranti avvocati che, dopo un lungo percorso di studi e dopo aver concluso nella maggior parte dei casi un periodo di praticantato con spirito di sacrificio e abnegazione, hanno proseguito la propria preparazione al fine di realizzare il proprio sogno. Nel frattempo, la disciplina transitoria, che prevede una modalità celere e semplificata nello svolgimento dell'esame, ha previsto la possibilità di espletarlo con tempi ridotti. D'altro canto, è sempre più importante anche la necessità di modificare la normativa vigente dell'esame da avvocato del 2012) in cui, accanto a una frequenza obbligatoria di corsi di formazione, potrebbero essere previste misure diverse e alternative, in modo da non pregiudicare l'effettivo esercizio della pratica. Questa proposta di legge può costituire il primo passo verso il cambiamento della normativa vigente sull'esame da avvocato, sempre più urgente. Su richiesta del Ministero della giustizia il Comitato tecnico-scientifico ha espresso parere sfavorevole in merito alla possibilità di svolgere le prove scritte secondo le ordinarie modalità, a causa dell'elevato rischio di contagio a cui sarebbero sottoposti i candidati. Stante l'impossibilità di un ulteriore rinvio dell'esame, che causerebbe una sovrapposizione con l'esame da avvocato 2021, è stato deciso di prevedere solo per la sessione 2020 un'ulteriore prova in sostituzione dell'ordinaria prova scritta. Tale prova, propedeutica alla seconda, avrà per oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta dal candidato tra materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo. Sarà svolta necessariamente in modalità di collegamento da remoto. Nello specifico, il candidato sarà presente nella sede d'esame: gli uffici giudiziari della Corte d'appello o i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, che potrà appartenere a qualsiasi pubblica amministrazione, purché dotato di laurea. La seconda prova avrà la durata di non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato, e sarà svolta a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima. avrà invece luogo davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e viene stabilita la facoltatività del collegamento da remoto. strumenti e modalità che aiuteranno a prevenire il rischio dei contagi, a tutela del supremo bene della salute. Tale misura è stata adottata per rispondere a questo difficile momento, con la speranza che di questo periodo possa rimanere solo un ricordo. Non possiamo permettere che le difficoltà ci sovrastino, ma dobbiamo piuttosto far sì che queste difficoltà possano rappresentare un'opportunità di cambiamento volta al miglioramento per il nostro Paese e per la nostra giustizia, una giustizia

Signor Presidente, onorevole sottosegretario Sisto, colleghi, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento che nasce in un momento emergenziale particolarissimo. Siamo sostanzialmente in un periodo bellico contro un nemico invisibile, in cui anche i giovani praticanti

un grande contributo per il funzionamento della stessa attività forense. Ci troviamo quindi a discutere un provvedimento a mio avviso è l'unico che in questa fase particolare possiamo approvare. Certo, non c'è più l'esame scritto, con le famose sette ore in cui

esame, molti anni fa come tanti che interverranno dopo o sono intervenuti prima di me, la selezione si era già verificata all'università. Ricordo ancora il primo giorno quando in aula magna, in un'atmosfera quasi surreale per un ragazzo che arrivava dalle scuole, mi ritrovai con tutti i professori schierati, allora eravamo in 630, e un professore disse di guardarci intorno perché solamente uno su quattro di noi sarebbe riuscito a laurearsi. Aveva sbagliato per difetto, perché in realtà su 630 ci laureammo in 100.

Pertanto c'era chi tentava di andare altrove per affrontare questo esame. Abbiamo avuto anche altri momenti, che forse qualcuno rammenta per il ricordo che è stato trasmesso: mi riferisco a quelli durante la guerra, quando si ritornava dal fronte, si davano gli esami e la cosa che si faceva un po' rocambolescamente era mettere la rivoltella - sono episodi veri - sulla cattedra, si prendeva il famoso voto e lo si portava a casa. Oggi siamo invece di fronte a una prova diversa, in cui dobbiamo selezionare 26.000 ragazzi. Tutti conosciamo l'apprensione, le difficoltà;

che cambiano dal giorno alla notte a seconda che si riesca a diventare avvocati oppure no. Pertanto, con molta delicatezza, in questo momento particolare in cui l'Italia ha vissuto una situazione davvero drammatica, a mio avviso dobbiamo guardare anche con occhio benevolo, con quello del

veramente consono, anzi, direi quasi naturale alla professione, quindi facciamo attenzione perché proprio questo tipo di esperienza potrebbe diventare un punto di riferimento anche per il nuovo esame, quando la situazione verrà considerata normale.

Signor Presidente, Piero Calamandrei diceva che gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto. La giustizia è una cosa seria. Sempre il grande giurista soleva dire: «Che vuol dire "grande avvocato"? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni». alla quale mi onoro di appartenere è una professione nobile, una professione che affonda le sue radici - io direi - nei primordi dell'umanità, da quando chiunque fosse sotto attacco o chiunque volesse far valere i propri diritti ha sentito la necessità di avere accanto a sé una persona preparata, capace di sostenerlo: *advocatus,* chiamato accanto a sé. Non è un mistero che negli ultimi tempi ci siano forti tentativi di sminuire la dignità di questa nobilissima professione cui apparteneva Marco Tullio Cicerone; professione che ha dato in tutto il mondo esponenti politici, statisti, persone che hanno saputo portare avanti i diritti umani. Una persona notissima - che nessuno sa facesse l'avvocato, per esempio - era il *mahatma* Gandhi. Oggi siamo di fronte a una modifica normativa - che speriamo tutti sia transitoria e temporanea, e che così resti - che ha visto comprimere in modo esasperato le facoltà dell'avvocatura. Negli scorsi mesi l'emergenza ha compresso notevolmente anche la dignità dell'esercizio della professione forense.

come all'umiliazione di partecipare a udienze nelle quali si può essere silenziati con un semplice *click* sul computer. Speriamo che tutto questo presto sia superato, che sia cancellato e che si possa tornare alla normalità dell'esercizio di una professione che deve poter mantenere la sua preziosa dignità.

Non sono certamente un fautore della chiusura alle giovani generazioni, ma non possiamo sottacere la necessità di garantire che il criterio per entrare a far parte della professione forense sia quello del merito

perché è vero che si è cercato - e diamo atto al Ministero e al Governo - di garantire i criteri di selettività, ma è anche vero che, come che sia, non siamo certo ai livelli garantiti, dall'esame nella sua forma ordinaria. L'avvocato deve saper scrivere

che l'emergenza che stiamo vivendo impone quest'anno di fare gli esami in maniera un po' anomala. Ho già sottolineato quali sono, a mio parere,

Questo metodo di valutazione mi lascia molto perplesso, perché si potrebbero verificare delle disparità

Ovviamente il tempo a disposizione è troppo breve, pertanto mi riservo di tornare su questi temi in fase di dichiarazione di voto. Avevo presentato anche un emendamento per fare in modo che i quesiti venissero scelti in maniera differente, ma poi si è deciso diversamente: trasformerò comunque l'emendamento in un ordine del giorno. Ci tengo anche a sottolineare che

Signor Presidente, com'è stato detto, siamo qui per garantire a dei giovani l'accesso alla professione.

e, come Partito Democratico, rivendichiamo una particolare attenzione a questi lavoratori della conoscenza. Nella precedente legislatura abbiamo ridotto da due anni a diciotto mesi il periodo di pratica, proprio per facilitare l'ingresso in questo particolare mondo del lavoro, diventato più irto di difficoltà e con condizioni lavorative e di reddito particolarmente pesanti.

di questi giovani nell'ufficio per il processo e questo è un modo moderno e intelligente di affrontare il tema del funzionamento della giustizia, del contributo dei saperi e anche della contaminazione delle esperienze.

patrocinio e questo innanzitutto per i destinatari, i cittadini non abbienti, ma anche perché è una forma di lavoro che interessa soprattutto i giovani. Recentemente ci siamo molto battuti affinché fossero sbloccate delle risorse per il pagamento di questi onorari, che sappiamo hanno un ritardo storico. Pensiamo che ancor più che contributi *una tantum* indiscriminati per i professionisti, in questo caso per gli avvocati, siccome i giovani sono i più esposti e siccome si tratta di lavoro effettivamente svolto e di oneri che lo Stato deve a questi lavoratori,

solo nelle corone di alloro, che possono sconfinare nella retorica. Abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare questo testo esattamente in questa direzione, direzione, pur misurandoci e cercando di tener conto dell'urgenza del provvedimento. Una questione che vogliamo affrontare è quella della trasparenza della prova d'esame per garantire non solo la genuinità, ma l'efficacia della prova stessa, o meglio per tutelare l'esito di questa prova che si svolge con modalità eccezionali, ma che richiederà e richiede anche l'impiego di risorse eccezionali, con un aumento delle commissioni che devono lavorare. C'è uno sforzo eccezionale da parte dello Stato ed è uno sforzo che va tutelato. Quindi chiediamo che, ove lo chieda il candidato, la prova possa essere videoregistrata. Vorrei Vorrei sottolineare che oggi la tecnologia offre una quantità di opzioni a costo zero, tant'è che ciascuno di noi può ormai - ahimè, dico io - registrare e videoregistrare qualsiasi cosa. Credo che siamo nelle condizioni di farlo e che la tecnologia possa e debba essere impiegata. L'abbiamo usata e la stiamo usando molto in epoca di Covid, quindi si può fare. La seconda questione è garantire la parità di trattamento, in questa forma eccezionale, diversa e sconosciuta, nella tempistica dell'apertura delle buste e dei quesiti; parità di trattamento per tutti coloro che devono affrontare questo esame. La terza questione riguarda gli studenti

concludere con due brevi osservazioni. Quando parliamo di accesso alla professione e di tutela della preparazione, quando studiamo le modalità che riguardano la professione dell'avvocato, parliamo sempre e comunque di garantire al meglio il diritto di difesa, che non è un principio

questo diritto di difesa deve essere ancor più garantito, perché in una società che cambia ci può essere la compressione e lo stravolgimento di diritti fondamentali in ogni campo; quindi la funzione dell'avvocato è ancora importantissima. Ma - attenzione - noi sappiamo che anche questa professione si deve misurare con la modernità; la sfida che dobbiamo accogliere che la modernità sia un'opportunità e non la trasformazione dell'ennesimo diritto

dell'accesso ad una professione, che misura la competenza e la preparazione, stiamo parlando di lavoratori della conoscenza. I lavoratori della conoscenza sono importantissimi proprio in questo mondo che cambia, che uscirà diverso dalla pandemia, che dovrà affrontare sfide che impegnano la conoscenza e la competenza e che non mettono più confini tra tecnologia e scienza da un lato e

e contaminare; io credo che ci sia un interesse sociale da parte di tutti affinché l'avvocatura sia all'altezza di questo compito e venga valorizzata per il valore sociale che ha e che riveste.

onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, è trascorso un anno dal *lockdown* totale che ha cambiato le nostre vite. È trascorso un anno esatto dalla mia interrogazione al ministro Bonafede, nella quale chiedevo se ritenesse di assumere iniziative urgenti per l'abolizione della prima prova scritta dell'esame di avvocato, procedendo direttamente alla seconda prova orale. è il 16 aprile 2020. Fui la prima a lanciare il grido d'allarme che proveniva da 26.000 praticanti, che chiedevano attenzione e di poter svolgere l'esame di abilitazione alla professione con modalità diverse, visto che la pandemia poneva ostacoli. Per questo motivo, ho usato tutti gli strumenti che i regolamenti parlamentari mi consentivano per sollecitare il precedente Governo, in particolare l'allora Ministro della giustizia, onorevole Bonafede, affinché venisse in Parlamento a spiegare perché 26.000 aspiranti avvocati dovessero essere sospesi in un limbo senza tempo, in attesa che l'epidemia da Covid-19 si placasse, in modo da consentire una anacronistica "tre giorni" di prove scritte. Al ministro Cartabia, per il tramite del sottosegretario Sisto, va il merito di essere stata tempestiva. Dopo aver affrontato, evidentemente, la problematica, si è resa subito conto che un esame che coinvolge numerosissimi candidati non poteva assolutamente essere svolto con le prassi consolidate, non in tempo di Covid-19: no, non sarebbe stato possibile. Quindi, mi complimento con lei

Un vecchio detto recita: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire; e nonostante le voci, quelle dal di dentro e quelle dal di fuori, si è continuato ad insistere sull'esame scritto, che avrebbe dovuto vedere migliaia di praticanti ospitati in grandi sale, per ben otto ore consecutive, ovviamente con grossi rischio di contagio. Grazie, quindi, ancora una volta al Ministro, che ha scongiurato questo rischio. Le siamo tutti molto grati. Ho presentato personalmente, come dicevo, una interrogazione parlamentare al ministro Bonafede, per spronarlo sull'emergenza che il totale indecisionismo sul punto aveva procurato. Ho tentato di sensibilizzare il precedente Governo affinché adottasse una soluzione che riconoscesse ai praticanti avvocati, così come era stato per ogni altra categoria professionale, il diritto di potersi abilitare mediante un esame orale, alternativo allo scritto, ma altrettanto serio e selettivo. In questo ultimo anno, ho avuto modo di ascoltare le esigenze e le richieste dei praticanti, tutte connotate da buon senso. Mi sono immedesimata nelle loro attese e quindi ho auspicato che si trovassero soluzioni per porre fine alle loro preoccupazioni. Essi rappresentano il futuro del nostro Paese e per troppo tempo sono stati lasciati in balia di un destino incerto. Oggi, finalmente, è giunto il momento, qui in Parlamento, di dare attenzione e di assumerci le nostre responsabilità per dare un meritato e degno futuro a circa 26.000 giovani aspiranti avvocati. Mi duole, però, dire che probabilmente si poteva fare anche qualcosa di più. Ho presentato più di un emendamento: uno, però, andava proprio in questo senso.

avrebbe, infatti, consentito un'accelerazione nei tempi e un minore dispendio organizzativo. Si sarebbe evitato di perdere ulteriore tempo prezioso, perché tanto sappiamo tutti che l'esame orale è una prova pubblica, in cui l'identità del candidato non può essere sicuramente sicuramente celata. Bisognava avere maggiore fiducia nella serietà dell'operato dei commissari chiamati a svolgere questo delicato compito. Sarebbe stato, a mio avviso, ragionevole una concentrazione dell'esame innanzi ad un'unica commissione; ancora, sarebbe stato meglio aumentare il termine dilatorio a trenta giorni dalla comunicazione al candidato e l'effettivo svolgimento della prova. In questo modo, si sarebbe potuto consentire al candidato sia di avere una maggiore preparazione specifica sia una maggiore organizzazione rispetto ad eventuali impegni lavorativi. Non dimentichiamo, infatti, che i praticanti avvocati, per poter vivere, devono anche lavorare. Trovo inoltre ingiusto che un praticante che venga esaminato su una materia durante la prima prova debba essere ancora testato sulla stessa nella seconda prova orale e, al contempo, obbligarlo a portare anche un'altra materia sostanziale. Se un praticante ha svolto una pratica forense solo in materia civile ed ha fatto la prima prova orale in diritto civile, perché mai deve essere esaminato, durante la seconda prova, sia sul diritto civile sia sul diritto penale? È un paradosso, che avrebbe meritato più attenzione ed una maggiore aderenza alla realtà. Mi rivolgo al senatore Urraro, con il quale ho avuto modo di interfacciarmi e che ho ringraziato per la sua grande disponibilità: saranno stati i tempi, evidentemente, e mi auguro che si possa fare meglio in futuro. Sarebbe stato più corretto garantire una coerenza ed una valorizzazione del percorso specialistico di pratica svolto da ciascun candidato; sarebbe stato meglio eliminare questo assurdo vincolo. Tuttavia c'è un fatto forse ancora più grave relativo all'esame, così come oggi è congegnato. L'attuale struttura, infatti, lascia un margine di discrezionalità troppo ampio alle singole sottocommissioni in ordine ai quesiti pratici della prima prova scritta. Il mondo dei

e che questi fossero trasmessi ad ogni corte d'appello ed estratti a sorte. In questo modo avremmo avuto quesiti uniformi su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, un metro di valutazione molto più ampio. Mi auguro che non si creino difficoltà con questo modo inoltre, che non ci si fermi a questo decreto-legge e che non torni tutto come era precedentemente all'emergenza Covid-19. Proprio per questo, in quest'ultimo anno ho intessuto rapporti, raccolto istanze e ascoltato le voci dei praticanti: non sono nuova nell'argomentare la questione dei praticanti avvocati. Ho presentato presentato anche una mia proposta di legge per riordinare l'*iter* dell'esame, perché è chiaro a tutti che l'esame necessita di essere riformato, per dare serenità nell'approccio al mondo del lavoro ai giovani praticanti avvocati. È inutile che ci prendiamo in giro: l'esame, così com'è strutturato attualmente, non è assolutamente meritocratico e non è in linea con quanto succede negli altri Paesi europei e non. Ad esempio in Spagna e negli Stati Uniti è previsto l'accesso alla professione forense con modalità molto più rapide e oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità di esame discendono ancora da un regio decreto del 1933. Questo determina una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extracomunitari, avendo così meno possibilità di esprimersi e di eccellere nel mercato del lavoro. Una riforma dell'esame di Stato è ormai assolutamente urgente, non solo perché anche a questi giovani laureati deve essere applicato il principio della libera circolazione dei servizi in Europa (una delle quattro libertà su cui si basa il mercato europeo comune), ma anche perché, soprattutto nel progetto di ricostruzione del Paese dopo la cessazione della pandemia da Covid-19, è fondamentale che i giovani possano dare il loro prezioso contributo e che ci sia il giusto ricambio generazionale della classe dirigente. Per cui, dopo l'approvazione del provvedimento odierno, mi auguro sia giunto il momento di prendere provvedimenti seri e pensati, di dare esaustiva risposta alla necessità di rendere di nuovo efficace e meritocratica la selezione attraverso l'esame di Stato, ormai troppo vecchio per adempiere ai suoi compiti. Chiaramente ho avuto modo di argomentare la mia proposta di legge in vari *webinar*; c'è stata la comparazione con altre proposte provenienti da altri partiti e ci sono state critiche, ovviamente, come sempre succede. Il mio auspicio è che si incardinino queste proposte di legge e si discuta confrontandosi, per addivenire ad una nuova legge, più snella, più praticabile, più adatta ai tempi. L'obiettivo che mi ero prefissata nella mia proposta di legge non era quello di escludere forme di valutazione definite al ribasso o di semplificare le procedure, ma di adattarle alla fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando da mesi. Non ritenevo e non ritengo che i *quiz*, come prova di esame, fossero umilianti per un aspirante avvocato, come è stato sostenuto. I *quiz* potevano

dovranno dimostrare anche una solida esperienza acquisita sul campo, ovvero nelle aule dei tribunali e nella redazione degli atti nelle cancellerie, per gli adempimenti. Orientarsi di fronte a un caso pratico, valorizzando quindi la pratica davvero svolta, deve essere la misura per selezionare legali di qualità, all'altezza della sfida professionale. Siamo consapevoli che la riformulazione delle prove di esame per l'esercizio della professione forense sia comunque contingente alla situazione di emergenza e che possa rappresentare una occasione per raccogliere criticità ed aspetti positivi che potrebbero essere valorizzati formulando, una volta superata la pandemia, una nuova prova di esame più al passo con i tempi, anche ipotizzando *stage* presso le cancellerie dei tribunali o

con cui, nella sostanza, aveva deciso di dare un'indicazione specifica di quelli che erano i suoi sentimenti, già espressi peraltro in vari scritti e discorsi. Mentre tutti noi aspettavamo di capire cosa volesse fare

della giustizia di Forza Italia, che ho l'onore di avere qui adesso come Sottosegretario, proprio perché esisteva ed esiste questo tipo di problema. Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e credo che l'altro segnale importante di carattere generale che fornisce l'interpretazione della linea del Governo il fatto che si cerca in tutti i modi di cominciare a sbloccare tutto quello che è concorso. Ad esempio stiamo discutendo oggi dell'esame di abilitazione degli avvocati;

anche con riferimento a tutti i concorsi pubblici che sono stati fermati dalla pandemia. Voglio sottolinearlo per un motivo: è vero che abbiamo un'Italia depressa perché le riaperture sono ancora lontane, ma è anche vero che la compagine ministeriale sta comunque lavorando per cercare di ritornare alla normalità e l'esame di abilitazione da avvocato o l'avvio dei concorsi hanno questa

magari vuole fare l'avvocato penalista e quindi battersi nelle aule contro l'accusa, oppure chi ama il civile ed è più portato allo scritto. Il titolo abilitativo oggi è fondamentale per chiunque voglia avere accesso a numerose professioni, perché è un supporto.

Moltissimi avvocati non svolgono in realtà la professione, ma magari fanno gli amministratori di sostegno, oppure si occupano delle procedure per l'esdebitazione o il sovraindebitamento, oppure lavorano in grandi studi di affari, quindi magari non vanno in aula, ma studiano i casi. La professione è cambiata moltissimo e ha sicuramente una serie ha sicuramente una serie di sfaccettature. Pertanto, consentire ai ragazzi oggi di avere questo titolo, pure in una situazione complessa come quella della pandemia, che giustifica un esame senza la parte scritta, è un segno di attenzione per chi vuole guardare avanti e trovare determinate soluzioni lavorative.

prudenti e attenti, sapendo cogliere le innovazioni importanti derivanti dalla pandemia, ma sapendo soprattutto guardare alla professionalità che deve avere chi affronta questo esame per avere un titolo

fino a tardi per consentire all'Assemblea di discutere il provvedimento e il Sottosegretario, perché pur non essendo un provvedimento perfetto, ma perfettibile come tutti, comunque segna un punto che è quello di cui vi dicevo prima: prima: il Governo ha cominciato a lavorare per riaprire i concorsi e ritornare lentamente e gradatamente alla normalità. *(Applausi)*. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

e che ha portato a dover decidere, in via emergenziale, come svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense. Non possiamo tacere il fatto che, all'interno della Commissione giustizia, già nei mesi scorsi con il precedente Governo e con il ministro Bonafede in particolare, abbiamo sollecitato più e più volte

ma mai nessuna risposta è giunta. Mai nessuna risposta è arrivata alla Commissione; sono state spedite delle lettere e delle richieste di audizione, ma mai nulla. Da questo punto di vista devo ringraziare il ministro Cartabia e il sottosegretario Sisto,

Sì, avremmo potuto fare una scelta, quella di far saltare l'annualità e non concedere la possibilità agli iscritti di quest'anno di fare l'esame, proprio in virtù dell'emergenza, però questo - lo sappiamo benissimo - avrebbe probabilmente creato maggiori problemi, maggiori ricorsi e criticità. Quindi si è arrivati alla scelta di trovare una soluzione diversa da quella dell'esame scritto. Sappiamo benissimo come funziona lo svolgimento degli scritti. Personalmente ho fatto l'esame a Milano, che si svolge in Fiera, tra migliaia di partecipanti,

insomma, le soluzioni possibili erano molte e la discussione sul punto è stata varia. Certo è che, se il predecessore del Ministro avesse ascoltato un po' di più, probabilmente in questo momento avremmo magari altre soluzioni, ma tant'è.

- siano responsabilizzate. Da un lato, dovranno essere consce di questa situazione emergenziale e, dall'altro, dobbiamo evitare che questo si trasformi in una maxi-sanatoria, come dicevo in precedenza. Abbiamo visto nelle settimane e nei mesi scorsi

è importante, ma non basta che l'avvocato sia menzionato all'interno della Costituzione. Il ruolo dell'avvocato dev'essere pienamente valorizzato e dev'essere di merito e concreto.

particolarmente importante, perché è il primo portatore della garanzia dei diritti del piccolo cittadino, quello del paesino o della signora anziana che ha una problematica con la bolletta della luce, perché gliene è arrivata una da 20.000 euro per un problema al contatore.

fondamentale. Ho svolto tale professione non perché sono figlio di avvocato, ma perché credevo fermamente nel suo ruolo. Quando ho iniziato a fare la pratica forense, mi sono insediato all'interno di uno studio

e noi di questo compito di tutela dobbiamo farci carico, perché, se non portiamo avanti i veri obiettivi,

togliamo un tassello tra il tribunale e il cittadino e, così facendo, eliminiamo la tutela dei diritti di tutti i cittadini. Mi auguro che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi questa discussione prosegua seriamente, in Commissione e in Aula, per far sì che quello della giustizia ritorni a essere un settore importante e fondamentale, com'è giusto che sia.

a poco più di un anno dallo scoppio della pandemia siamo tutti consapevoli della grave situazione che il Covid-19 ci costringe ad affrontare. Per sconfiggere questo tremendo nemico invisibile, sono state molte le decisioni difficili che la politica ha dovuto prendere, con l'aiuto dei tecnici e della comunità scientifica. Ciononostante, l'emergenza purtroppo non è ancora alle spalle. Il numero dei contagi non ci permette di tirare un sospiro di sollievo e ci obbliga a mettere in campo tutti gli strumenti in nostro possesso per evitare un aggravio. Per i medesimi motivi, in autunno, per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale, è stato deciso il rinvio della prova scritta dell'esame di Stato per diventare avvocato. Tale prova, tradizionalmente svolta nel mese di dicembre, era stata differita alle date 13, 14 e 15 aprile prossimo venturo, nella speranza che nel frattempo il contesto sanitario fosse migliorato. Tuttavia, ad oggi non vi è stato il miglioramento auspicato e appare ancora impensabile svolgere le prove scritte secondo le modalità classiche. È infatti noto che lo svolgimento della prima prova dell'esame da avvocato richiede almeno tre giorni di tempo, raggruppando migliaia di candidati in varie sedi sul territorio nazionale. Con uno sguardo alle esperienze degli anni passati, ci accorgiamo che sarebbe complicato e troppo gravoso rispettare la normativa vigente in tema di assembramenti, la quale non consente di raggruppare più di trenta persone in un'unica sede. I candidati che ogni anno sostengono contemporaneamente la prova scritta per diventare avvocato sono infatti alcune migliaia e solitamente sono dislocati in padiglioni fiera o strutture equivalenti. Risulta impensabile raggruppare oggi così tante persone in un unico luogo. Allo stesso modo, Allo stesso modo, appare molto complicato pensare di dividere agevolmente i candidati in piccoli gruppi senza dover sostenere costi organizzativi elevatissimi, anche solo in termini di personale necessario per il controllo del corretto svolgimento delle prove. Il rischio di contagi, inoltre, resterebbe ugualmente troppo elevato: si pensi ad esempio all'attività preliminare obbligatoria del controllo dei codici o al consumo degli alimenti durante le prove scritte, che durano almeno sette ore. Il comitato scientifico a cui il Ministero della giustizia ha richiesto un parere si è così espresso, senza lasciare spazio ad alcun dubbio: considerando l'andamento epidemiologico e tenuto conto delle modalità di svolgimento delle prove, non è pensabile svolgere in sicurezza l'esame scritto di abilitazione alla professione forense. Nemmeno un rinvio ulteriore degli scritti risolverebbe il problema, a causa dei lunghi tempi necessari per le correzioni e per il successivo esame orale. Finirebbe quindi per accavallarsi alla sessione di abilitazione Ancora più impensabile appare l'ipotesi di non svolgere l'esame di Stato 2020, innanzitutto perché vorrebbe dire mortificare le aspettative future di oltre 26.000 persone che hanno presentato domanda in quell'anno. Sarebbe infatti inaccettabile vanificare gli sforzi di tutti coloro che, dopo il lungo percorso di studi in giurisprudenza, hanno concluso il periodo di praticantato, spesso devo dire senza alcuna retribuzione, investendo risorse personali e delle proprie famiglie. Il loro sacrificio e la dedizione che hanno dimostrato meritano tutto il nostro rispetto e il nostro impegno, affinché sia posta in essere una soluzione per garantire loro l'accesso alla professione di avvocato. Inoltre, vorrebbe dire arrendersi al virus e dimostrarsi inermi in questa che è una vera e propria guerra. Per questi motivi si è scelto d'intervenire normativamente per sostituire, solo nella sessione 2020, la prova scritta con un'ulteriore prova orale. Tale prima prova, propedeutica alla seconda, avrà ad oggetto un quesito pratico applicativo nella formula della soluzione di un caso che richieda competenze di diritto sostanziale e processuale. Il candidato potrà scegliere tra le materie di diritto civile, penale o amministrativo, in linea con la tradizionale tradizionale scelta del parere e dell'atto previsti dalla prova scritta. Il tempo assegnato sarà di un'ora dalla fine della dettatura del quesito. Il candidato avrà a disposizione i codici commentati con la giurisprudenza per la prima mezz'ora; al fine dell'esame preliminare del quesito, e gli verranno restituiti

Il candidato potrà prendere appunti, che non saranno oggetto di valutazione. Esaurita la discussione, la commissione si riunirà in camera di consiglio, comunicando al candidato l'esito della prova. La prima prova orale sarà svolta dinanzi a una commissione diversa da quella della corte d'appello di appartenenza del candidato. La scelta della commissione sarà effettuata secondo le modalità tradizionali di sorteggio, Il candidato dovrà presenziare presso gli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di appartenenza o presso i locali del consiglio dell'ordine, alla presenza del segretario di seduta, che ne controllerà il corretto svolgimento, svolgimento, mentre la commissione esaminatrice sarà necessariamente collegata da remoto. La seconda prova si svolgerà invece in presenza, dinanzi alla commissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e avrà una durata minima di quarantacinque minuti e massima di minuti e massima di sessanta. In tal modo si ritiene che si ridurranno al minimo i rischi di diffusione del contagio, tutelando allo stesso tempo aspiranti avvocati e commissari giudicanti. La tecnologia ci viene in soccorso, permettendoci di ripensare le nostre abitudini, senza rinunciare a momenti indispensabili come la selezione

Pensiamo a una riforma dell'ordinamento professionale forense che l'avvocatura ha atteso per oltre ottant'anni, perché prima era regolamentata da un regio decreto-legge del 1933. Nel 2012 abbiamo ottenuto una regolamentazione dell'avvocatura

mattina. La delicatezza delle prove a cui si accingono 26.000 aspiranti avvocati rappresenta qualcosa di significativo in un momento di compressione dei diritti. Lo dico sempre: prima prima ancora che difendere i diritti dei cittadini a cura dell'avvocatura, qui bisogna custodirli da parte di chi oggi racchiude e verifica tante patologie sociali e tante istanze grezze di giustizia che devono essere trasformate in domanda di giustizia intesa quale bene comune. Gli interventi che si sono susseguiti sono significativi e hanno tracciato un *excursus* anche storico dell'intera sequenza, nel corso degli anni, dell'accesso alla professione forense, che merita sicuramente un'attenzione *ad hoc* in un momento successivo a questa fase epidemiologica da cui ci auguriamo di uscire davvero

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.2, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3).

Invito alla trasformazione in ordine del giorno

impegna il Governo: a valutare la possibilità in sede attuativa che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale,

previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati, esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato».

affinché ai candidati che superano la prima prova, anziché trenta giorni, ne vengano concessi sessanta, prima dell'inizio della seconda. Vorrei ricordare che

(almeno colui che sapeva di averne svolta una con buone probabilità di superarla) aveva tutto il tempo per preparare le materie da presentare a quella orale. Nel nostro caso, abbiamo una prima prova orale che tiene luogo di quella scritta. Sarebbe quindi ragionevole lasciare un lasso di tempo

di questo provvedimento, ma certamente questo aiuta i candidati che già devono affrontare una situazione molto difficile, come del resto tante altre categorie e, insomma, lascia il tempo per poter studiare le materie che saranno oggetto di esame nella seconda prova.

per il fatto che vi sono delle grandi difficoltà organizzative, in un anno orribile quale quello corrente, per poter raggiungere gli obiettivi proposti che, anche a livello di impegno del Governo, in questo momento non posso assolutamente assumere. Non me ne vorranno i colleghi, ma anche sugli ordini del giorno il parere è quindi contrario.

che volevano corsie preferenziali per le vaccinazioni. Bravi gli avvocati, male i magistrati.

Non c'è alcuna difficoltà a prendere atto che l'esigenza manifestata con l'ordine del giorno sia indubbiamente legittima.

Inviterei, ove i proponenti fossero d'accordo, al ritiro degli ordini del giorno, con l'intesa che in sede propria e opportuna si possa riconsiderare logisticamente l'esigenza manifestata.

Riprendo il ragionamento che ho fatto in discussione generale. È un provvedimento che sicuramente è stato leggermente migliorato, ma che ancora presenta delle criticità che mi auguro, in sede di decreto ministeriale, siano superate. Certamente non si può fare a meno di osservare che i criteri valutativi non saranno sicuramente omogenei

dicevo, è auspicabile che in sede di decreto ministeriale vengano indicati dei criteri valutativi per le singole commissioni in maniera tale da assicurare quella parità di trattamento e di valutazione che oggettivamente nel provvedimento in esame non esiste, proprio per le modalità ivi previste. Pur rendendoci conto che stiamo parlando di un di un esame che si svolgerà in siffatta maniera soltanto per quest'anno, a causa - come ho già detto in precedenza - della situazione di emergenza sanitaria, è necessario assicurare

quel che è accaduto con le tariffe forensi, con l'eliminazione dei minimi, a mio parere ha provocato un grossissimo danno alla categoria, che vive un momento di grandissima difficoltà. È innegabile che molti studi hanno dovuto chiudere e molti avvocati svolgono la loro attività da casa, non avendo la possibilità economica di tenere uno studio aperto. In questo senso è auspicabile che ci sia una selezione vera e che possano accedere alla professione solo le persone realmente preparate e vivono nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata la loro attività. Spero anche che in sede di decreto ministeriale venga superato il problema della formulazione dei quesiti. Abbiamo presentato un ordine del giorno che prevede che i quesiti vengano predisposti poco prima della prova stessa ed estratti a sorte davanti al candidato, che peraltro si trova in remoto, nel senso che verrà esaminato da una commissione che si trova altrove, mediante i consueti programmi Zoom, Skype o simili. questo non consentirà di adottare un criterio omogeneo, perché i quesiti potranno essere diversi da sede in sede e potranno anche avere un'oggettiva differenza di difficoltà.

A questo punto, nei criteri di valutazione, bisognerà quindi badare a che il candidato effettivamente si presenti come capace di ragionare, manifesti la conoscenza quantomeno dell'istituto nei suoi principi fondamentali e in qualche modo

non potesse poi ripresentarla all'esame orale. Ormai ci si sta avviando verso la specializzazione degli avvocati - personalmente non sono mai stato d'accordo,

anche la modifica delle modalità di svolgimento della pratica forense. Oggettivamente è difficile che oggi la pratica prepari in maniera seria allo svolgimento della professione.

andare sul campo e verificare direttamente nelle aule giudiziarie lo svolgimento di un processo. Tutto verrebbe molto più facile e soprattutto gli studenti sarebbero molto più formati per lo svolgimento di quella che decideranno essere la loro professione.

stamattina in Aula, di migliorare il testo su quelle che ci sembravano alcune criticità. Alcune nostre proposte sono state accolte e di questo ringrazio il relatore e il Governo. Altre invece sono state respinte, con varie motivazioni. Ciononostante, riteniamo che comunque questo sia un atto dovuto nei confronti degli oltre 26.000 giovani aspiranti professionisti, che hanno svolto il loro *curriculum* di studio e la pratica e hanno dunque il diritto di essere valutati per l'accesso alla professione. Siamo convinti che ciò che oggi decidiamo sia una misura straordinaria, dettata dalla grave situazione pandemica che sta attraversando l'Italia e non solo. Si tratta di una situazione straordinaria che certamente non potrà diventare la regola, perché nel provvedimento ci sono delle criticità insormontabili. Nel momento in cui non si può svolgere una prova scritta,

coinvolgono migliaia e migliaia di candidati (3.000-4.000, nelle sedi più grandi). È chiaro che, senza una preselezione scritta, basarsi unicamente su una prova orale è certamente difficile. Noi ci rendiamo conto che la situazione straordinaria non poteva portare ad altra soluzione che a quella in esame, e semmai ci rammarichiamo

su alcuni aspetti rimane, e ne facevano cenno anche altri colleghi prima di me, in particolare - mi rivolgo al Governo, perché in sede di decreto di attuazione ne tenga conto - riguardo alla omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale

a una selezione seria, oggettiva e uniforme su tutto il territorio nazionale: ciò che le regole che stiamo provando non ci garantiscono. Anche l'idea

si basano per poter formulare le domande ai candidati, secondo me deve essere seriamente presa in considerazione, proprio per evitare i quesiti fai da te che a quel punto potrebbero contenere tutto e il contrario di

Come già hanno sottolineato molti colleghi - poi hanno ritirato tutti gli emendamenti, perché hanno trovato una posizione contraria da parte del Governo - già la durata della prima prova

di saper ragionare sul diritto e sulla materia, oltre che conoscerla. Un conto è conoscere la nozione, altro conto è saper ragionare intorno

potrebbero oggettivamente essere pochi, anche se vengono calcolati dal momento in cui il quesito è posto. Forse sarebbe stato più opportuno prevedere un termine maggiore, non tanto per la risposta (mezz'ora può andare benissimo), quanto per lasciare un po' più di tempo al candidato per l'approfondimento e per l'esame attraverso i codici commentati con la giurisprudenza, attraverso

perché stiamo parlando di una professione di rilievo costituzionale; stiamo parlando di avvocati, e cioè di professionisti ai quali i cittadini devono affidare la tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, che si tratti di di penale o di civile. Pensiamo davvero, signor Sottosegretario, di poter valutare la capacità professionale dei candidati

anche in condizioni eccezionali sia garantita la massima serietà possibile alla prova e, con tempi così rigidi e predefiniti, certamente credo che

si giunga così in ritardo a trovare una soluzione, esprimiamo il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame, perché ribadisco ancora una volta

che pone fine - questa è la cosa più importante - a una situazione di incertezza che riguarda concretamente la vita professionale e le prospettive di 26.000 persone

Lo facciamo - ripeto - lanciando un messaggio positivo che le istituzioni unitariamente, superando anche le divisioni e le differenze, mettono al primo posto: la necessità di rispondere a quell'esigenza, a quel bisogno che tanti ragazzi e tante ragazze ci hanno manifestato negli ultimi mesi. Il decreto-legge interviene in emergenza e tale va considerato. Questo provvedimento si spiega solo perché vogliamo rendere possibile l'esame di Stato per

il provvedimento ha il merito di consentire lo svolgimento degli esami mantenendo uno *standard* di serietà e di rigore

una carriera difficile ma - come è stato detto da molti - affascinante come quella dell'avvocato. Credo che la doppia prova orale, così come concepita, costituisca il sistema più convincente da mettere in campo per coniugare la garanzia di un esame realmente probante con i limiti di un esame che, a causa della pandemia, si deve fare da remoto. da remoto. In questi mesi, non solo i parlamentari che si occupano di giustizia ma tanti altri,

su come rendere rigoroso il sistema di definizione e scelta dei quesiti che saranno alla base delle prime prove orali. Ebbene,

tanti quesiti quanti sono gli esaminandi del giorno, per poi scegliere tra gli stessi quesiti, mi pare una buona Forse si poteva fare di meglio, ma questa mi pare una buona soluzione che garantisce trasparenza e serietà. È un ordine del giorno: ci aspettiamo

a garanzia di tutti - di videoregistrare il proprio esame, essendo un esame che viene fatto da remoto ed essendo i sistemi operativi predisposti per le registrazioni. Anche in guardiamo con favore all'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo presentato al riguardo e ci auguriamo che eventuali problemi tecnici possano essere superati. Penso infatti che il tema della videoregistrazione, che peraltro ci è stato posto da tanti

abbiamo accolto positivamente l'emendamento del relatore che consente di non escludere dalla seconda prova orale la materia che è stata scelta

l'emendamento del relatore raccoglie le sollecitazioni venute da diversi di noi.

Per queste ragioni e per il lavoro fatto in tempi brevissimi, voteremo a favore di un provvedimento utile,

un passaggio a livello che ne blocca alcuni) sia un tema fondamentale da riprendere nei prossimi mesi.

Presidente, onorevoli colleghi, la pandemia ha ridefinito molti aspetti della nostra vita sociale e, per evidenti ragioni legate all'elevata probabilità di diffusione del virus in luoghi molto affollati, ha avuto effetti anche sullo svolgimento dei concorsi pubblici, tra cui quello di abilitazione alla professione forense. un esame molto atteso ogni anno da migliaia di aspiranti avvocati e che quest'anno, per la precisione, ha coinvolto circa 26.000 persone. Per la prima volta dal Dopoguerra, infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato. Com'è emerso anche dalla relazione tecnica, il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al Comitato tecnico-scientifico, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale, non sia possibile l'esecuzione in sicurezza delle prove scritte in considerazione, appunto, dell'andamento epidemiologico. Le prove scritte dell'esame 2020, che si dovevano svolgere ad aprile 2021, avrebbero inoltre imposto un ulteriore differimento, con l'impossibilità di portare a termine la correzione degli scritti ed effettuare quindi gli orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione. La forma del decreto-legge è stata necessaria, non solo perché sorretta dai motivi di urgenza legati alla pandemia, ma anche perché imposta dalla natura primaria delle norme cui occorre derogare, che tuttora disciplinano l'esame da avvocato. Com'è noto, l'esame da avvocato tradizionalmente consta di tre prove scritte e di una prova orale, tutte prove che hanno la medesima finalità, quella di testare la capacità del candidato di saper argomentare un caso giuridico. Le nuove prove, invece, consistono in due esami orali. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dei commissari che effettueranno gli esami, viene stabilito che la prima prova orale, che ha natura preselettiva, consiste nell'esame di un caso pratico, la cui soluzione viene esposta dinanzi a una commissione diversa da quella insediata presso una sede di appartenenza - che a sua volta è diversa da quella del candidato - e individuata mediante sorteggio. Per rendere meno difficoltosa tale prova, assolutamente nuova e per la quale i candidati potrebbero non essere preparati, il Governo si è impegnato a fornire a chiarimento delle esemplificazioni. Inoltre, attraverso un emendamento del relatore approvato all'unanimità dalla Commissione, si consentirà al candidato di poter estendere la seconda prova orale anche alla materia già scelta per la prima prova. La *ratio* del decreto è dunque quella di preservare la salute dei candidati e dei commissari di esame e garantire, al contempo, una certa qualità nella selezione sostituisce ben tre prove scritte - fondata sulla capacità, indispensabile per chi si approccia alla professione, di argomentazione e soluzione di un quesito giuridico. Altre modalità di esame richieste da più parti, come ad esempio i quiz a correzione informatizzata, sarebbero state senz'altro più semplici forse avrebbero messo ancora di più al riparo dai rischi di metri di valutazione diversi da parte delle numerose commissioni diversamente composte, ma certamente non sarebbero state altrettanto efficaci a testare la capacità giuridico-argomentativa degli aspiranti, perché sarebbero state una mera analisi della preparazione nozionistica, affidata inoltre alla velocità delle risposte. Un bravo avvocato, oltre ad una solida preparazione, deve sapersi orientare tra norme, dottrina e giurisprudenza ed avere buone doti espositive. L'avvocato è infatti un attore fondamentale nel processo; è il professionista del foro delegato ad assistere e difendere una parte in un giudizio civile, penale, amministrativo, tributario, un ruolo che, se esercitato bene, non solo garantisce un diritto costituzionale come il diritto di difesa, ma può anche dare un notevole contributo ad una decisione giusta. Del resto per un buon avvocato non è indispensabile possedere l'*ars oratoria*, l'arte di parlare in pubblico; non c'è bisogno di essere un sofista come Gorgia o un avvocato come Cicerone, ma è sufficiente saper convincere il giudice sulla giustezza delle proprie tesi ed essere utile e affidabile per il proprio cliente. Certamente un avvocato deve anche saper scrivere, lo sappiamo. Ma ritengo che le nuove e temporanee modalità di esame, seppur diverse dal solito, possano essere idonee in questa fase e costituiscano un corretto bilanciamento tra necessità di selezione dei candidati da abilitare e tutela della salute, assolutamente giustificata dall'emergenza che stiamo vivendo. Quindi in bocca al lupo a tutti coloro che aspettano questo momento. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali.

storicamente, tra le libere professioni, quella dell'avvocato ha avuto sempre una disciplina particolare. Solo negli anni successivi, di recente quasi, la libera professione di dottore commercialista si è uniformata al sistema di selezione dell'avvocato.

basti pensare che nel Dopoguerra l'avvocato era soltanto colui che aiutava a garantire il diritto di difesa nelle cause. Riflettendo a lungo - come il sottosegretario Sisto ricorderà - nella discussione sulla previsione dell'avvocato in Costituzione, io in Costituzione, io ho valorizzato quell'aspetto dell'avvocato a cui faceva riferimento Emanuele Pellegrini. A cosa mi riferisco? Nella congerie delle leggi, enorme nel nostro sistema, non tutti i cittadini hanno la possibilità di rendersi conto dei propri diritti e dei propri doveri. Quindi la capacità dell'avvocato di rendere edotto il cittadino dei propri diritti e doveri ne fa un un consulente privilegiato, anzi direi il garante dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. *(Applausi)*. Prendete in considerazione qual è il principio dell'eguaglianza, la quale si verifica soltanto se io e un altro cittadino abbiamo la stessa capacità e la stessa possibilità di conoscenza di quali sono i nostri doveri e i nostri diritti; e questo lo rende possibile soltanto un avvocato. Quale avvocato? Un avvocato professionalmente preparato e adeguato. sono nato in Campania e quindi la mia prima esperienza è stata quella di entrare nella reggia di Castel Capuano, dove erano allocati gli uffici giudiziari della Campania (tribunale, corte d'appello). C'è una grande sala, il cosiddetto Salone dei busti, dove ci sono i busti marmorei non dei magistrati,

la presenza dell'avvocatura all'interno della società. La società era tale che mi ha insegnato questa esperienza. Io ricordo sempre operai e contadini che, nel momento in cui c'erano i grandi processi in corte d'assise, andavano ad assistere al processo. «Che facciamo stamattina? Andiamo ad assistere al processo». Adesso non c'è più questa usanza; eppure era una grande usanza di comprensione di quelle che erano le valutazioni. Devo dire con molta tristezza che però già allora, in molti di quegli ambienti, si diceva: «*quann' parl' o fetent'?*» (che era il pubblico ministero).

giusto che, proprio per questa ragione, sia stato mantenuto per anni un sistema di accesso all'avvocatura completamente diverso dalle altre libere professioni. Tutti voi sapete, che un medico e un ingegnere, nonostante siano responsabili della nostra salute, della stabilità dei ponti e delle nostre case, fanno soltanto un esame di abilitazione, sei mesi dopo la laurea, all'interno della stessa facoltà universitaria. Agli avvocati, no, non basta la laurea in giurisprudenza. Occorre, invece, un praticantato di due anni e poi, finalmente, l'esame. Esame che, nel tempo, è diventato più un concorso che un esame. Un tempo era un esame di verifica dell'abilitazione e della capacità dell'avvocato, delle sue capacità, capacità, non solo difensive, ma della sua conoscenza e modalità di rapportarsi alla legge e al cittadino che gli chiedeva un parere. Per cui, di fatto, l'esame era, più che altro, una verifica degli elementi minimi e c'era l'idea che la professione avrebbe fatto, poi, l'avvocato. Oggi, invece, assistiamo a una selezione quasi concorsuale, che è derivata non dalla necessità delle leggi o dalla necessità connessa a una difficoltà maggiore della professione, ma semplicemente dal numero di partecipanti, compreso quello di chi parteciperà al prossimo concorso, pari a 25.000 candidati. Voi vi rendete conto

una modalità che ripartisce nello stesso modo, come era tra gli scritti e gli orali, due modalità di prove. Una prima prova, sia pure orale, ma che è, né più né meno, quello cui facevo riferimento anche prima: prospettare prospettare un quesito e che il candidato abbia la capacità e la possibilità di esprimersi e di dare conto della sua preparazione. Molti sono

si è discusso a lungo, in Commissione, sull'opportunità di stabilire un tempo massimo e un tempo minimo dell'esame. Anch'io sarei stato più favorevole - e l'ho rappresentato al Sottosegretario ad individuare solo un tempo minimo di durata, perché il tempo massimo è difficile da individuare. Tuttavia, una volta individuato il tempo

la domanda, è talmente evidente che il candidato non sa nulla perché risponde malissimo, non c'è necessità di proseguire per mezz'ora o tre quarti d'ora. Bisogna avere la capacità di essere degli interrogatori: chi fa l'interrogazione deve avere una preparazione per comprendere il candidato, così come avviene in tutte le università. Per questa ragione, con i limiti e con le correzioni che sono state apportate, signor Sottosegretario, noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Ci auguriamo,

rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, l'epidemia di coronavirus ha sorpreso e messo in ginocchio il mondo intero. Nessuno l'ha scelta o desiderata, semplicemente c'è e con essa tutti noi siamo chiamati a fare i conti. A causa di questa pandemia ogni settore della società umana è costretto a ridimensionare le proprie aspettative, a modificare gli stili di vita e i progetti, a patire danni di tipo economico, talvolta, lo sappiamo bene, insopportabili. Fra questi c'è anche il settore della giustizia, che, fra mille difficoltà, ha cercato di dare risposte nei tribunali e negli uffici preposti alle immutate esigenze delle nostre comunità. Ricordiamo chi si è trovato a dirigere gli uffici: i magistrati, il personale e gli avvocati, spesso - troppo spesso - lasciati soli, con protocolli diversi nei diversi territori, che hanno creato solo confusione. Il provvedimento su cui oggi dobbiamo esprimere il nostro parere viene alla luce nello stesso contesto emergenziale e si pone di fronte a quest'Assemblea con prepotente urgenza. Avrebbe potuto essere licenziato prima, magari dal precedente Esecutivo? Lascio a voi questa risposta e soprattutto evito di cedere alla tentazione della polemica. Ma certo, se oggi siamo qui, è perché il nuovo Governo ha scelto di affrontare con responsabilità e pragmatismo le difficoltà di questa stagione. A proposito, voglio anche ringraziare i componenti della Commissione che presiedo, che nella trattazione di questo decreto-legge hanno dimostrato la medesima responsabilità e una grande capacità di sintesi e di collaborazione e hanno consentito di concludere rapidamente e bene l'*iter* previsto. Ciò dimostra che il lavoro parlamentare non rappresenta una perdita di tempo e che, anche nelle urgenze, lo strumento del decreto-legge si rivela efficace e, nello specifico, migliore di qualsiasi Un ringraziamento va anche ai rappresentanti degli ordini professionali che abbiamo audito in Commissione e di cui, quando possibile, abbiamo raccolto i contributi. Da loro, come sempre, ci aspettiamo una vigile collaborazione. Presidente, anche io sono avvocato e ricordo, come molti colleghi, la trepidazione con cui ho affrontato, ormai qualche anno fa, l'esame di abilitazione alla professione forense. Un esame non facile, capace di garantire la preparazione dei candidati, perché, quando saranno chiamati ad esercitare la loro funzione, dovranno farlo con l'equilibrio e la professionalità che il loro prezioso ruolo richiede. Anche questo nuovo esame, che i tanti candidati attendono da dicembre scorso, dovrà garantire la medesima preparazione, con regole e modalità eccezionali - certo - ma senza facilitazioni, senza aiuti, senza sconti, perché non possono e non devono esistere avvocati di serie B e avvocati di serie A. Ripercorrendo il testo del decreto-legge che ci accingiamo a votare e anche la gran parte degli interventi di chi mi ha preceduto, posso affermare che sì, quella che stiamo dando oggi è la risposta migliore possibile di fronte alle esigenze presenti; contemperare quindi la salvaguardia della salute e dell'ordinato svolgimento delle prove con l'esigenza di garantire i livelli di preparazione e di merito. Merito: ripetiamo ancora questa parola perché il Paese mai come oggi ne ha bisogno. Colleghi, avremmo potuto rassegnarci a un'ulteriore proroga, scegliere di non decidere, di non esprimerci, di rinunciare alla nostra funzione, ma avremmo fatto il male della giustizia e avremmo mancato di lealtà nei confronti delle donne e degli uomini che attendono risposte e che sono, anche loro, vittime di questa pandemia. Per tale ragione dico di guardare al futuro consentire attraverso il nostro voto ai tanti praticanti in attesa di risposte di misurare la loro preparazione e di mettersi a disposizione della giustizia.

Affrontate il vostro esame senza timori. La pandemia ha cambiato il mondo, non cambierà però i valori della civiltà umana: credibilità e merito nella professione forense, come in tutti gli ambiti della vita, vinceranno sempre e faranno la differenza.

è un decreto di emergenza. Nonostante infatti l'avvio della campagna vaccinale, la diffusione della malattia da coronavirus non si è attenuata e poiché le prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, per la prima volta dal dopoguerra, non si sono potute tenere, esse sono state rimandate al 13, 14 e 15 aprile 2021. Tuttavia l'attuale gravissima situazione epidemiologica impedisce ancora una volta lo svolgimento delle prove scritte. Pertanto il Governo, in accordo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni giustizia del Senato e della Camera ringrazio anche il sottosegretario Sisto - sentito il Comitato tecnico scientifico, ha cercato la migliore soluzione possibile, pur sapendo di non accontentare tutti. Ciò al fine di evitare i contagi soprattutto tra candidati e commissari. Si è dovuto tener conto della necessità di evitare assembramenti e spostamenti nel territorio nazionale di circa 26.000 praticanti avvocati e di circa 500 addetti ai lavori tra magistrati, avvocati e personale amministrativo. Si è altresì dovuto tener conto dell'impossibilità di svolgere le tre canoniche prove scritte in diverse sedi del territorio nazionale. Pertanto si è dovuto pensare a diverse soluzioni logiche organizzative affinché questi giovani avvocati praticanti possano al più presto entrare nel mondo del lavoro, ma in tutta sicurezza. Nessuno infatti può essere lasciato indietro. Si è dovuto anche tener conto dell'impossibilità di portare a termine la correzione di eventuali prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento anche della sessione di esame 2021. È questo infatti il motivo per cui non si è accolto l'emendamento del senatore Balboni, che avrebbe voluto ampliare il termine dalla fine della prima prova orale alla seconda. Ebbene, colleghi, in questo quadro abbiamo deciso di abbandonare l'ipotesi delle prove scritte in presenza e sostituirle con una prova orale a carattere preselettivo, cioè propedeutica rispetto alla canonica prova orale. Si tratta di un vero e proprio orale rafforzato. Il primo orale dell'esame consiste nella discussione di una questione pratica applicativa nella forma della soluzione di un caso in materia a scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo. La sottocommissione predispone tre quesiti per ogni candidato per la materia prescelta e li colloca all'interno di buste distinte e numerate, tra le quali il candidato ne sceglierà una. Il tempo per lo svolgimento sarà di sessanta minuti. Dispiace non aver potuto accontentare i giovani avvocati che chiedevano maggiore tempo, magari giustamente; si tratta comunque di trenta minuti per esaminare il quesito e di trenta minuti per la discussione, sempre con la possibilità di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato. Conclusa la prova, la commissione si ritirerà in Camera di consiglio per la valutazione e l'esito sarà comunicato subito dopo. La seconda prova orale pubblica dovrà svolgersi, come ho detto prima, entro trenta giorni dalla prima e questo perché si spera di concludere la prima parte dell'esame a settembre e la seconda parte entro novembre, proprio per riuscire a fare anche la sessione di esame di avvocato di dicembre 2021. La discussione verterà su cinque materie scelte preventivamente dal candidato con l'aggiunta del codice deontologico. A questo proposito voglio ricordare anche l'emendamento, approvato ieri sera in Commissione e votato oggi in Aula, per cui si è data ai praticanti avvocati la possibilità di scegliere tra la materia del diritto civile o del diritto penale, anche se tale materia è già stata scelta per il primo orale. Riguardo alla disciplina delle sottocommissioni, stante il maggior numero di candidati, la normativa prevede che siano composte da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti devono essere avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, mentre gli altri possono essere magistrati, anche militari, professori universitari o ricercatori, fermo restando che il presidente deve essere sempre un avvocato. In merito al reperimento del personale amministrativo necessario per la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e sottocommissioni, in deroga alla legge del 2012, si estende tale funzione anche al personale amministrativo in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di almeno una laurea triennale. Il problema invece degli spazi idonei a consentire lo svolgimento della prova di esame viene risolto chiamando a turno i candidati presso gli uffici giudiziari e consigli dell'ordine ove hanno la residenza e si svolge con il collegamento da remoto con la commissione, che sarà diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, ossia individuata per sorteggio e ciò al fine proprio di rispettare tutte le misure relative all'emergenza sanitaria. Per la seconda prova orale è prevista invece la facoltà, non più l'obbligo, del collegamento da remoto. Dispiace anche qua che non sia passato l'emendamento che avrebbe consentito ai praticanti avvocati residenti all'estero di sostenere l'esame presso i consolati o le ambasciate della Repubblica italiana. *(Applausi)*. Invece, in caso di positività al virus, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere, con istanza corredata da adeguata prova documentale sanitaria, di fissare una nuova data per la prova e questo anche in caso di malattia, sempre grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle. Voglio concludere, Presidente, anticipando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento, ma anche facendo una considerazione doverosa. Questa è sicuramente una prova di esame eccezionale per i futuri candidati alla professione di avvocato, perché anche loro sono stati pregiudicati dal coronavirus e da questa pandemia. Nonostante tutto hanno continuato a studiare, continuano a crederci e vogliono entrare anche loro nel mondo del lavoro. Tuttavia, come dicevo, è una prova eccezionale, perché la classe forense deve rimanere una categoria seria e qualificata e ciò nell'interesse sociale di tutti i cittadini che fanno affidamento sulla giustizia per la tutela dei loro diritti.

Desidero innanzitutto ringraziare l'Assemblea. È la prima volta che prendo la parola su un provvedimento legislativo e il caso ha voluto che fosse sulla prova di ammissione per gli avvocati: se ci avessi provato, non ci sarei riuscito. Sono molto grato alla Commissione, che ha consentito un risultato rapido efficiente, nell'interesse dei nostri 26.000 ragazzi, che tutti hanno ricordato. Vorrei soltanto rammentare come le competenze possono significare anche efficienza e questo mi piace segnalarlo. Il dialogo serve e anche su provvedimenti di questa rilevanza si può incontrare quella sinergia, che rende l'attuale momento del Parlamento italiano estremamente positivo ed utile.

l'episodio più grave dai tempi della guerra fredda. Mi riferisco all'arresto di un ufficiale della Marina italiana, che è stato fermato insieme a un militare russo, per spionaggio. Si tratta di una grave minaccia alla sicurezza dello Stato, che dimostra che anche l'Italia è coinvolta nella strategia di offensiva russa. Dopo le campagne di disinformazione lanciate da organi vicini al Cremlino, per condizionare la politica italiana, questo episodio dimostra che il livello dello scontro si sta alzando ulteriormente. Signor Presidente, visto che il Copasir è paralizzato dal fatto che la sua composizione e la sua presidenza non corrispondono a quanto dettato dalla legge, il Gruppo Fratelli d'Italia chiede che venga immediatamente in Assemblea a riferire il Presidente del Consiglio o, per lui, il Sottosegretario con la delega ai Servizi. *(Applausi)*.

Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, restituiamo oggi all'esame dell'Assemblea un documento molto importante per noi e per le prossime generazioni, che tiene insieme visione e proposte, valori e progetti. Il lavoro delle Commissioni riunite 14a e 5a, così come avvenuto per le linee guida, è stato impegnativo, con l'aggravio questa volta di essere dovuti passare attraverso le maglie di una crisi di Governo che ci ha visti attendere la definizione dei nuovi interlocutori per procedere all'analisi e all'esame del Piano. Abbiamo operato dando seguito a un articolato ciclo di audizioni che ci ha permesso di maturare i contenuti di questo documento che riporta, a mio avviso, una sintesi equilibrata delle diverse sensibilità che animano il nostro Parlamento, non solo nell'ampia maggioranza. Come relatore, unitamente avverto l'esigenza di utilizzare il tempo a mia disposizione per mettere in evidenza alcuni punti del documento, a valle di una coordinata ripartizione col collega Pesco. Inizio da due aspetti che definisco di sistema. Il primo riguarda la necessità di trasformare le politiche per i giovani, attualmente indicate come priorità trasversali nelle varie missioni, in un pilastro specifico e autonomo, come peraltro previsto nel regolamento UE del 18 febbraio. Si tratta di una scelta che condividiamo nella sua *ratio* perché coerente con le finalità stesse di questo Piano, che è per l'appunto rivolto alle nuove generazioni. L'altro punto di sistema che intendo portare all'attenzione dell'Assemblea è invece più specifico e riguarda la necessità perentoria di scongiurare il rischio che, in nome della tempistica stringente e dei criteri altrettanto esigenti che il Piano porta con sé,

diventasse l'ostacolo alla progettualità nei settori e nei territori dove i divari sono maggiori e dove è più urgente la necessità di andare a operare una perequazione. Non possiamo in alcun modo permettere che i criteri stringenti in ambito tempistico fungano, tra la beffa e una sorta di contrappeso, da ulteriore leva che finisca in sostanza per ampliare quel divario per il quale siamo destinatari di questa mole di risorse e in ragione del quale stiamo attuando il Piano in esame. Sarebbe un corto circuito imperdonabile, che decreterebbe nell'immediato e senza appello il fallimento di quella che è un'iniziativa storica che ci offre l'Unione europea. Scontiamo infatti da anni una disomogeneità in servizi e infrastrutture materiali e immateriali che la pandemia ha solo reso più evidenti, rispetto alla quale, tuttavia, oggi abbiamo l'opportunità di operare. Per Per questo, parità di genere, giovani e sviluppo del Mezzogiorno sono alla base della nostra attenzione e corrono lungo tutto il Piano. Su questi tre elementi trasversali non possiamo in alcun modo fallire. Rispetto al primo - la parità di genere - è a tutti chiaro come la crisi che ancora oggi attraversiamo si è abbattuta con particolare ferocia sulle donne e sulle donne lavoratrici. Abbiamo tutti letto i dati, che fanno rabbrividire: i dati sull'incidenza della loro espulsione dal lavoro nel 2020, a cui si vanno a sommare ulteriori gravami, quali sono i costi di gestire i figli in DAD, di continuare a dare assistenza nel contesto familiare, ad esempio, ai genitori anziani e, non da ultimo, anche dell'eventuale convivenza con la violenza nella propria casa. Abbiamo di conseguenza deciso di indicare chiaramente al Governo un set importante di impegni per cominciare praticamente a recuperare quello che fotografiamo come un *gap*, ma che per profondità, complessità ed interconnessione è un universo che nel nostro Paese necessita di una vera e propria energica iniziativa multisettoriale. Di qui l'impegno

così come l'impegno nel superamento della disparità nei servizi educativi, che aleggia su tutto il nostro territorio, l'aumento dei congedi di paternità, la revisione del sistema del servizio di cura degli anziani e la promozione dell'accesso alle facoltà STEM, incrociando quindi strategie per il presente e investimenti per il futuro. Anche in ambito economico sono tanti gli strumenti e le misure che presentiamo oggi nel documento all'esame dell'Assemblea: dal mero punto di vista funzionale, con la previsione a livello burocratico della comunicazione *once only*, alla riforma della pubblica amministrazione, così come di quella fiscale, per passare poi agli incentivi alla digitalizzazione delle imprese o - ancora a una serie di puntuali indirizzi per una delle migliori espressioni del *made in Italy,* quale è appunto il sistema della moda Italia, che intende anch'esso sviluppare il suo impegno nell'ambito del *green* e della sostenibilità. Infine, in questo mio serratissimo periplo di relazione da affidare all'Assemblea (per i cui contenuti rimando totalmente al documento depositato e distribuito), mi permetto di dedicare un ultimo passaggio al Mezzogiorno, perché è la ragione per la quale riceviamo più risorse di altri Paesi e non è certamente un merito, né un vanto. Può piacere o meno, ma l'Unione europea destina al nostro Paese il 25 per cento complessivo dell'ammontare di risorse del Next generation EU in vista di tre parametri,

Proprio per tale ragione, la percentuale totale delle risorse e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza non dovrà in alcun modo essere pari o inferiore al 34 per cento per il Sud, come prevede la norma ordinaria, quanto tale percentuale legata alla popolazione è bastevole a mantenere il *gap* e non a ridurlo. Abbiamo l'esigenza di rimettere insieme i pezzi di un'Italia a oggi spaccata, marciano con ritmi, mezzi e strumenti a volte insopportabilmente diversi e disomogenei. Il documento arricchisce e istruisce il Piano iniziale con una certa dose di dettagli che oggettivamente mancavano nella versione approvata a gennaio. Abbiamo operato in modo da meglio definire le parti eccessivamente timide e dare maggiore visione e campo a quelle che si presentavano in modo incomprensibilmente limitato. Faccio riferimento, ad esempio, alla necessità che l'Alta velocità colleghi tutta l'Italia, tutta la dorsale adriatica e tutta la dorsale tirrenica della Penisola (dico tutta perché da qui si misura un fatto di civiltà). Mi riferisco, come altro esempio, alla centralità del Mediterraneo per lo sviluppo del sistema portuale che non può, né deve continuare a essere declinato secondo solo i due porti *hub* di Genova e Trieste.

È allora evidente che non possiamo aderire alla *vision* che inquadra i porti di Taranto e Augusta - cito due esempi - in una logica di resistenza rispetto a quelli delle altre sponde del Mediterraneo e secondo un piglio di vocazione essenzialmente turistica, perché in Italia

con la pandemia si è reso evidente come il patrimonio di potenzialità inespresse del nostro Paese sia ampio. Faccio riferimento alla sinergia, tutta da costruire, data dal turismo *slow*, da quello *green* e dall'incontro con le proposte tipiche agroalimentari italiane (elementi che abbiamo messo bene a fuoco nel documento). Chiusa questa digressione e riprendendo il tema del Mezzogiorno, chiediamo interventi puntuali anche per le zone pienamente operative. Infatti, se procediamo alla realizzazione delle infrastrutture in quell'esagono, dobbiamo poi operare di conseguenza per permettere loro di funzionare. Concludo, signor Presidente, e lo faccio aprendo un'altra breve parentesi.

Chiedo quindi al Governo una presa di impegno forte e condivisa nel predisporre, di pari passo con la realizzazione del Piano, un programma di ridestinazione di queste risorse a favore di progetti che non rientrano negli stringenti requisiti del regolamento UE/2021/241, ma che rispondono invece a precisi interessi nazionali di sviluppo come, ad esempio, l'ammodernamento della rete stradale e autostradale anche nel Sud del Paese. modo, dati i tempi concitati, bisogna pensare a procedure normative *ad hoc* per garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR. Consegno dunque al Governo queste mie riflessioni,

di approvazione definitiva e di monitoraggio di quanto accadrà dopo l'invio del Piano a Bruxelles.

purtroppo non abbiamo elementi significativi di dettaglio per capire se il Piano che si sta perfezionando con il dialogo con l'Unione europea effettivamente tenga conto delle cose che avevamo indicato nel precedente passaggio in Aula: questo sfortunatamente lascia ancora qualche elemento di non

fare il possibile per ricomprendere la tutela degli ecosistemi tra gli obiettivi che il Governo italiano si è dato attraverso la realizzazione del Piano. Abbiamo delle sacche e delle lacune ambientali veramente importanti. Mi riferisco

le acque interne, le cose vanno un pochino meglio, visto che arriviamo a 50 per cento di classificazione delle acque non buone con riferimento ai laghi. Per fortuna, le acque sotterranee che raggiungono lo stato buono superano il 50 per cento, arrivando al 57,6

ambientali che sono stati creati. Sempre sull'ambiente, c'è da fare sicuramente qualcosa in più a proposito di una delle misure che ha comunque spazio; mi riferisco al superbonus che stiamo realizzando in questi mesi in tutta Italia. Si dovrebbe fare di più per riuscire ad allungare il più possibile gli anni nei quali si potranno svolgere i lavori con l'aiuto pubblico. *(Applausi)*. Sappiamo che non è semplice, perché l'Europa ci chiede di riuscire a spendere queste risorse entro il 2026 e quindi il programma di assorbimento di questo credito fiscale andrebbe andrebbe più a lungo; però dobbiamo fare il possibile per cercare di allungare il superbonus almeno fino al 2023 e, chissà, magari anche oltre. È importante puntare molto sull'inclusione sociale. Purtroppo in Italia, in Italia, visto il periodo che stiamo vivendo, la situazione è veramente critica. Le associazioni che abbiamo sentito durante le audizioni ci hanno portato la testimonianza di molte persone in difficoltà; ci riferiamo alle persone sole, alle persone non autosufficienti, alle persone diversamente abili

in modo da rendere più semplice per queste persone l'accesso alle richieste e l'ottenimento dei servizi sociali. È una misura straordinariamente importante, che dobbiamo realizzare attraverso una riforma.

non è questo ciò che serve. Serve più personale per lo svolgimento di questi servizi, serve raggiungere personalmente questi pazienti, anche a domicilio, servono risorse umane in più. Sappiamo che il Piano non è finalizzato a questo, però potremmo studiare dei progetti, anche limitati nel tempo, che fungano da

popolazione che erano abituate a stare bene e che ora si sono impoverite. Sono veramente tante e molte sono legate al sistema produttivo. Quindi, bisogna trovare una soluzione che riesca a coniugare le esigenze del sistema produttivo e delle realtà più piccole, che sono veramente in difficoltà, con le famiglie di riferimento.

della banca che presta soldi alle persone in difficoltà sia ridotto. In questo modo, riusciremmo ad aiutare sia gli istituti di credito sia le persone, perché riceverebbero più risorse. È poi importante, per le famiglie legate a delle aziende in difficoltà, aziende che non riuscirebbero a ripartire neanche con l'aiuto economico, trovare sistemi più

facile la ripartenza di queste persone, attraverso strumenti che già esistono, come il codice della crisi d'impresa e la legge sul sovra indebitamento. È però necessario far dialogare questi strumenti, affinché una famiglia legata a una piccola impresa, che non ha trovato sviluppo e che purtroppo si arena in questo periodo, abbia la facoltà di capire qual è la miglior soluzione per uscire da una crisi debitoria e poter ripartire. È importante fare di più. Lo si è detto anche quando abbiamo discusso le linee guida: è una cosa fondamentale. Questo è un periodo particolare. Molte famiglie e molte aziende stanno male, ma dobbiamo ammettere che molte famiglie, legate magari a persone che non hanno problemi col lavoro, hanno accumulato in questo periodo più risparmio rispetto ai mesi precedenti. Sarebbe importante riuscire a far dialogare il risparmio accumulato con l'aiuto necessario per famiglie e imprese. Quindi, magari anche all'interno di questo Piano, visto che serve alla ripartenza, potremmo trovare strumenti adatti per riuscire a far dialogare questa possibilità di offerta con le necessità di persone e famiglie; nonché trovare gli strumenti utili per investimenti e aiuti alle piccole realtà e alle piccole imprese. Concludo, ringraziando ancora tutti per il lavoro fatto.

signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la Next generation EU è la grande occasione per lo sviluppo del nostro Paese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza può permettere all'Italia un vero cambio di rotta e un'importante accelerazione, rendendolo un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata, dinamica, ma, allo stesso tempo, con una vera rivoluzione e stabilizzazione della sua struttura sociale. È un piano di ripresa che non dovrà riportarci al tempo di prima, ma dovrà permettere di costruire un'Italia nuova, che sappia raccogliere le opportunità collegate alla tradizione ecologica e digitale, creando nuova occupazione, ma anche migliorando la qualità del lavoro e dei servizi, in particolare la struttura sanitaria e l'organizzazione del sistema scolastico-formativo. È un piano di resilienza, perché l'emergenza pandemica ed ecologica rende indispensabile prepararsi bene ad affrontare le complesse problematiche, già presenti, ma ulteriormente accentuate dalla pandemia, al fine di poter ripartire e preparare il futuro. Potremmo riassumere tutto ciò in una frase: governare le trasformazioni senza subirle. La proposta del PNRR prevede una strutturazione secondo i tre assi strategici che ben conosciamo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Inoltre, comprende un articolarsi con le sue sei missioni orizzontali, che mirano a raggiungere dei grandi obiettivi strategici, che potremmo definire essere destinati ad un riequilibrio sociale e ad un adeguato sviluppo culturale: la parità di genere; l'accrescimento delle competenze e delle prospettive di occupazione dei giovani; il riequilibrio territoriale, con particolare attenzione al Mezzogiorno. In particolare la missione salute, che, soprattutto in questo momento, rappresenta uno dei punti fondamentali del programma, comprende due principali campi su cui focalizzare l'attenzione, che dovranno permettere uno scatto positivo del nostro Sistema sanitario, con un graduale e progressivo miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, dell'assistenza sanitaria, cercando di colmare, oltretutto, le naturali differenze territoriali esistenti tra le varie zone del nostro Paese, raggiungendo una maggiore omogeneizzazione delle varie prestazioni erogate e dei servizi forniti, con un miglioramento della sua organizzazione strutturale, sia a livello territoriale che ospedaliero. Ecco quindi, in quest'ottica, da un lato, il previsto potenziamento dell'assistenza di prossimità territoriale e della telemedicina e, dall'altro, l'attenzione alla ricerca e alla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, che comprende, in particolare, il nuovo fascicolo sanitario. Tutta la rete territoriale, con la sua riorganizzazione, permetterà di curare meglio i pazienti, soprattutto quelli cronici, nel proprio domicilio, tra i loro affetti, riconoscendo l'importanza della componente psicologica nel complesso delle cure erogate. Tutto ciò si potrà realizzare con l'adeguata implementazione dell'assistenza domiciliare integrata con le case della comunità e, per le cure intermedie, negli ospedali di comunità. Fondamentale, inoltre, è il miglioramento della telemedicina, capace di abbattere le distanze e permettere collegamenti con le strutture specialistiche di riferimento. Tutto ciò permetterà una migliore gestione anche dell'acuto e di fornire assistenza in situazioni di emergenza, migliorando la qualità delle prestazioni domiciliari erogate. Si potrà e si dovrà fare meglio e rapidamente presso il letto del malato. Altro aspetto che vorrei sottolineare è la valorizzazione della ricerca, che non deve essere più considerata come una fonte di spesa, ma come un vero investimento per il futuro; non un ramo secco, in cui sprecare soldi pubblici, ma un punto fondamentale su cui investire per non arrivare sempre in ritardo alle grandi battaglie, come è appunto quella della pandemia. Vaccino anti-Covid *docet*. A tal proposito, occorre aumentare i fondi per la produzione dei vaccini anti-Covid e incrementare in Italia la produzione di dosi vaccinali su licenze di case farmaceutiche straniere. Secondo il MoVimento 5 Stelle la strada migliore per ottenere ciò rimane la sospensione temporanea dei brevetti. Non dimentichiamo mai che solo una vaccinazione globale permetterà il vero successo della campagna vaccinale. Più ricerca equivale a più occupazione, meno fuga di cervelli all'estero. Il nostro Paese deve diventare un soggetto attivo, svolgere una funzione trainante e di *leadership* nell'ambito dei consessi internazionali scientifici, così come da tradizione e per le altissime competenze e professionalità presenti nelle nostre università. Le maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nella realizzazione dei tanti progetti compresi nel Piano potrebbero, a mio avviso, riscontrarsi nel riuscire a realizzare i giusti equilibri, i corretti coordinamenti e gli adeguati collegamenti tra le diverse competenze e le strutture organizzative coinvolte, stante anche la massiccia mole di programmi e progetti da realizzare. Occorreranno competenze, professionalità, superamento di veti incrociati o di barriere, anche culturali, per non dire demagogiche, che spesso ostacolano e rallentano l'adeguato percorso realizzativo delle riforme e dei grandi progetti. Viviamo un momento storico impegnativo e difficile. È una sfida importante per l'Italia e per gli italiani; per poterla vincere occorre il contributo di tutti, ciascuno per la sua parte. Solo lavorando tutti assieme si riuscirà a superare questa crisi globale, sconfiggere la pandemia, ripartire con basi solide e con idee chiare e nuove, realizzando gli obiettivi previsti. *(Applausi)*.

onorevoli colleghi, membri del Governo, in risposta alle conseguenze dell'emergenza pandemica sull'economia, l'Unione europea ha riconosciuto la ricerca scientifica tra le priorità di investimento pubblico per il rilancio. È in questo ambito che vorrei portare il mio contributo oggi. Vorrei farlo affrontando quattro aspetti essenziali per la ricerca, che toccano la bozza del Piano nazionale Il primo aspetto riguarda le risorse per la ricerca. Poter contare, grazie a Next generation EU, su una quota maggiore di risorse può permetterci di colmare quel divario sul numero di dottorati di ricerca l'anno (9.000 in Italia contro i 15.000 in Francia e i 28.000 in Germania), o quello sul numero di ricercatori pubblici (appena 75.000 in Italia contro 110.000 in Francia e 160.000 in Germania). questo è quanto proposto dagli studiosi firmatari del cosiddetto Piano Amaldi, in parte recepito nella relazione delle Commissioni che oggi esaminiamo. Aumentare il numero dei ricercatori significa avere più idee in campo, più strade immaginate, un maggiore potenziale di innovazione a beneficio dell'economia nazionale e della competitività a livello internazionale. però perché questi traguardi non si raggiungono in automatico, perciò, mirando ad aumentare il numero di studiosi, dobbiamo chiederci cosa vogliamo offrire loro, come pensiamo di sviluppare le loro migliori idee per trasformarle in valore aggiunto, con quali strumenti vogliamo intercettare e valorizzare i talenti. Per quanto, al secondo punto del mio intervento, si trovano le misure per i giovani. Investire nei giovani significa una sola cosa: una sola cosa: garantire loro libertà di accesso ai fondi pubblici attraverso procedure competitive e valutazioni competenti e indipendenti delle loro proposte. È perciò un bene che nella bozza del PNRR sia previsto un programma di finanziamento pubblico pluriennale, e quindi duraturo, almeno per cinque anni, per accendere nuovi laboratori di ricerca, per far nascere nuovi *team* di ricerca che studino tutto - mi verrebbe da dire - tutto ciò che è utile sapere e saper fare, in ogni ambito umanistico e scientifico, guidati da giovani ricercatori. Dovrà essere un piano finalizzato a trovare e far emergere i talenti diffusi nel Paese e farne arrivare altri dall'estero, aprendo loro la strada per farli diventare le nuove eccellenze della ricerca internazionale del futuro. Un programma ambizioso, ispirato ai bandi del Consiglio europeo della ricerca, l'European research council (ERC), rivolti a ricercatori agli inizi della carriera. Un ERC italiano quindi a cui i giovani possano guardare con fiducia per collocarsi presso quegli enti pubblici che ne vorranno e sapranno accogliere progetto e indipendenza. Passo ora al terzo punto, per esprimere invece una forte preoccupazione sulla bozza del PNRR. La preoccupazione è legata al fatto che non possiamo compiere sempre gli stessi errori che poi costringono a complesse e difficili modifiche in corso. Nella bozza del PNRR vi è l'intenzione di introdurre nel già diffuso, complesso e sottofinanziato sistema della ricerca pubblica del Paese, altri sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo e altri venti campioni territoriali di ricerca e sviluppo - cioè altri 20 più sette centri di ricerca, o così si intende - verosimilmente iperfinanziati. Non se ne capisce la necessità o, meglio, non possiamo creare nuovi enti senza aver proceduto prima ad una approfondita analisi che dimostri la necessità di questi nuovi centri fisici che siano 20, 27 o solo sette nuove strutture, per capire anche come dovranno essere organizzati rispetto agli enti esistenti e ai tanti gruppi di ricerca teorica e applicata che nel Paese già svolgono esattamente le funzioni che verrebbero assegnate a questi nuovi enti. enti. È un'analisi necessaria, colleghi, oggi assente; necessaria anche a comprendere e spiegare ai cittadini in che modo i centri ipotizzati possano essere sostenibili, compatibili e complementari con gli enti - ben 135 - che già si occupano di ricerca nei vari settori. Una volta accertato questo, andrà individuata una procedura competitiva, aperta a singoli enti e gruppi di ricerca, in cui presentare progetti dettagliati e motivati per la realizzazione di tali strutture, per capire dove collocarli nel Paese e perché, affinché possano essere selezionate le migliori proposte di contenuti di quei centri, dalle migliori cordate di studiosi, i più rispondenti alle esigenze del territorio e della comunità. Per esempio, rispetto a uno dei sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo, il Centro nazionale per l'intelligenza artificiale, mi chiedo stato valutato il rischio di una sovrapposizione con enti e attività già esistenti, il rischio di spendere i fondi europei per una moltiplicazione inutile di enti. Da alcuni autorevoli studiosi del settore mi è stato segnalato che non risulta sia stata mai fatta un'analisi e una consultazione preventiva. Mi chiedo anche se il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica, che dal 2018 ha una specifica branca sull'intelligenza artificiale, sia stato interpellato: a me non risulta. Guardate, di eccellenze e talenti diffusi in tutto il territorio il nostro Paese è già ricco. istituzioni che fanno ricerca ogni giorno con l'obiettivo di creare nuove conoscenze utili alla crescita di imprese e territori, quindi del Paese, e che comprende università, ospedali di ricerca ed enti pubblici di ricerca, anche se il loro lavoro resta spesso sconosciuto a cittadini e rappresentanti politici. A guardare gli esiti dei lavori di questi studiosi, che già esistono, c'è di che essere orgogliosi; i nostri giovani si formano evidentemente bene, ma mi chiedo se tutto ciò sia noto. Mi chiedo ad esempio quanti, nelle istituzioni impegnate a disegnare il nostro futuro, siano a conoscenza del fatto che sono state le università di Modena e Reggio Emilia e il San Raffaele di Milano a sviluppare il primo farmaco nel mondo occidentale a base di staminali e che grazie alle staminali e a trent'anni di ricerca, sempre nei laboratori di Modena, si è riusciti a ricostruire la pelle di un bambino che ne aveva persa più dell'80 per cento a causa di una malattia rara, rendendogli una vita normale. Mi chiedo quanti sappiano che gli studiosi del CNR di Cagliari e dell'Università di Sassari sono numero uno al mondo sulla genomica; che l'Università Federico II di Napoli è conosciuta in tutto il mondo per gli studi sul rischio e la storia delle eruzioni del Vesuvio, oltre che per la robotica; che i geologi italiani sono al secondo posto al mondo, dietro gli Stati Uniti e davanti alla Cina, per gli studi sulle frane e al primo posto in assoluto nello studio delle grandi estinzioni biologiche; che sono italiani i ricercatori di astrofisica che hanno descritto per la prima volta i vortici ciclonici di Giove, grandi come la terra, che stazionano ai due poli del pianeta, una scoperta valsa la copertina di «Nature»; che all'università di Bologna si studia l'origine della scrittura e la linguistica delle lingue scomparse; che l'Università La Sapienza di Roma, proprio quest'anno, ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali grazie agli studiosi delle scienze dell'antichità. Mi chiedo se non sia proprio questa mancanza di conoscenza di ciò che già abbiamo il motivo per cui ciclicamente viene proposta la creazione di centri e strutture *ex novo*. Ma, attenzione, l'ignoranza di questa realtà non libera dalla responsabilità di decisioni improvvisate. Arrivo al mio quarto e ultimo punto con una riflessione, o meglio una proposta: credo che, oltre a non avventurarsi nella creazione di nuovi centri che non discendano da un'analisi della loro necessità, sia importante lavorare per valorizzare le eccellenze diffuse nel Paese. Esistono e sono intorno a noi, a partire dalle università e dagli enti di ricerca. Una strategia potrebbe prevedere azioni su base competitiva, riservate a università ed enti di ricerca, a partire da quelli delle zone più isolate del Paese, le cosiddette aree interne, fornendo un'arma in più contro fenomeni come il depauperamento demografico, sociale ed economico di quei territori. In concreto, si tratterebbe di emanare un bando, volto al finanziamento, ogni anno per cinque anni, di almeno 10-15 progetti, da 20 milioni di euro l'uno, sulla base di una valutazione aperta, competitiva e trasparente. Guardate che l'ordine di grandezza economico non è troppo dissimile da quanto ha fatto la Germania nel promuovere il programma della sua strategia di eccellenza. Non ha creato nuovi enti, ma ha aperto bandi e ha messo

Si potrebbe veramente fare così. Inoltre, adesso è forse giunto il momento di consentire l'accesso alle nuove risorse, assegnate sempre su base competitiva, a tutti i ricercatori, a qualsiasi ente appartengano, a prescindere quindi dagli steccati amministrativi di provenienza: già questa sarebbe una riforma semplice e rivoluzionaria. Innovare Innovare non significa per forza costruire da zero. L'innovazione più coraggiosa risiede spesso in un cambio di paradigma nella gestione delle risorse, in una riforma che che serve a valorizzare ricchezze ed eccellenze sconosciute o sottovalutate. La competitività del Paese passa anche da un rilancio omogeneo degli investimenti in ricerca pubblica, umanistica e scientifica, e da procedure aperte e trasparenti, libere e competitive. In conclusione, consapevole che il PNRR alla nostra attenzione è ancora in via di definizione, non posso che esprimere il mio giudizio positivo sul documento che il Senato sta licenziando, soprattutto quando afferma esplicitamente che debba essere prevista - e qui cito il documento - «una analisi preliminare dei bisogni, laddove nuove strutture», i centri di ricerca, «vadano ad integrare un contesto preesistente, così come si ritiene necessaria la definizione di criteri principi e metodi relativi alla gestione degli affidamenti, nonché l'individuazione del soggetto preposto alla selezione dei progetti da finanziare». indicazioni frutto di una ragionevolezza, che dovrebbe presiedere alla definizione di ogni politica pubblica e che mi auguro sentitamente che il Governo vorrà impegnarsi a recepire, affinché il nostro Paese possa beneficiare appieno, per il presente e per il futuro, della competizione ad armi pari tra le migliori idee, da qualunque parte d'Italia provengano.

il nostro Paese avrà a disposizione 209 miliardi di euro, a seguito della terribile pandemia che ancora stiamo vivendo. Si tratta di una risposta storica della Commissione europea alla crisi sanitaria, economica e sociale.

lo strumento finanziario si chiama Next generation EU non a caso, perché le politiche attuative dovranno essere in funzione del beneficio delle nuove generazioni. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha in sé questo obiettivo grande e ci consegna una enorme responsabilità. Alla sanità saranno destinati 20 miliardi, ancora insufficienti per gli obiettivi che ci poniamo; a mio avviso, dobbiamo investire tali risorse tali risorse mossi da una voce che, in cuor nostro, dovrà sempre dirci: mai più un sistema sanitario così impreparato alla pandemia, con sovraffollamento negli ospedali, con l'aver trascurato e penalizzato i pazienti di altre patologie (cardiopatici, malati di cancro, neurologici, pazienti affetti da malattie rare, che ancora oggi sono penalizzati), con una terra di nessuno sui territori e con una differenziazione così forte tra Regioni che stiamo vedendo

che deve prevedere al centro una sanità territoriale in cui non ci sia più un deserto tra medico di base ed ospedale. Il medico di base dovrebbe essere un primario territoriale di mettere insieme *équipe* multidisciplinari, specialisti sul territorio e continuità con gli ospedali. Occorre una sanità territoriale in grado di assistere a domicilio soprattutto gli anziani, i non autosufficienti, i pazienti cronici; una sanità di prevenzione con stili di vita corretti, di modo che i nostri giovani di oggi invecchieranno meglio; una sanità che metta al centro salute e ambiente: le parole del presidente Pesco sono state molto significative in questo senso. Quanto più ci prendiamo cura dell'ambiente, più ci prendiamo cura della nostra salute. È necessaria una sanità di prossimità che abbia strumenti decenti, degni di un Paese del mondo contemporaneo; una sanità di telemedicina, di digitalizzazione, che usi l'intelligenza artificiale in tutto il territorio nazionale. Il nostro Paese eccelle per esperienze di qualità, ma la sfida deve essere quella di far sì che tutto il territorio nazionale comprenda queste innovazioni importanti. Ripeto, la digitalizzazione, le cure personalizzate,

Ebbene, nell'attuale PNRR ci sono questi propositi, ma dobbiamo metterci ragione, anima e cuore per trasformare il nostro Sistema sanitario, per prepararci anche ad eventuali altre epidemie con proposte concrete, visione e progetti, come dicevano i nostri relatori. Un minuscolo virus ci ha dimostrato che se va in ginocchio la sanità, immediatamente va in crisi l'economia, il lavoro e la nostra intrinseca umanità, che è fatta di relazione con l'altro da sé, che ci è negato in questo momento, soprattutto per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. di ripresa e resilienza è la nostra sfida politica, etica e direi esistenziale. Aspettiamo che il Governo venga a discutere i progetti concreti con il Parlamento, perché è essenziale che noi rappresentanti della Nazione, come recita la nostra Costituzione, possiamo dare il dovuto contributo al citato Piano nazionale di resilienza, con le sue risorse. Noi politici dobbiamo essere in questo momento un tutt'uno con la cittadinanza. A noi classe politica

e ci impegnerà nei prossimi anni. Penso che il peso della responsabilità sia comune a tutti noi: provare ad immaginare un futuro, mai come in questo momento incerto, richiede un grande sforzo individuale e collettivo, localistico e globale, e ci impone inoltre di accettare allo stesso tempo una sfida per il futuro che implica la costruzione di un nuovo modo di vivere sulla nostra terra. Tutto questo nel bel mezzo di una pandemia. Il *green new deal,* il nuovo patto verde dell'Europa, europea sulla biodiversità per il 2030 hanno evidenziato già prima della pandemia il profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo. Vorrei sintetizzare questo concetto: ogni uomo dovrebbe portare con sé un albero con il quale scambiare vicendevolmente ossigeno e anidride carbonica per vivere.

La proposta del PNRR trascura completamente un tema fondamentale che riguarda tutte le missioni del Piano, ovvero la pianificazione dell'utilizzo dello spazio terrestre e marino che serve per la realizzazione delle infrastrutture da esso previste. Se non ci occuperemo al più presto di questo tema, creeremo conflitti sociali ed economici non facilmente gestibili. Oggi è il 31 marzo e il piano di utilizzo dello spazio marittimo avrebbe dovuto essere già operativo; senza di esso si rischia di danneggiare l'economia del mare. Temo che senza un piano condiviso con tutti i portatori di interesse rischieremo di favorire la transizione energetica a sfavore della pesca e del turismo. Lo spazio, però, ci serve anche per rigenerare il capitale naturale, il che significa tutelare la biodiversità degli ecosistemi naturali Tutti abbiamo accettato di incrementare almeno del 30 per cento le aree protette terrestri e marine, ma non mi sembra di aver letto da nessuna parte come ottemperare a questo impegno. Questo ci riconduce ancora alla pianificazione. Le nicchie ecologiche di pregio che consentono la rigenerazione del capitale naturale vanno individuate come primo elemento e solo dopo si potrà decidere dove e cosa costruire. Nel PNRR ci si è dimenticati che l'Italia è una penisola con più di 8.500 chilometri di costa, aree protette marine, arcipelaghi, isole abitate, porti e che dunque il mare e l'economia blu sono elementi fondamentali per il nostro Paese che vanno tutelati e promossi. I cambiamenti climatici *in primis* porteranno all'innalzamento del livello del mare, quindi alla scomparsa di buona parte delle nostre coste, con danni umani ed economici enormi. Il *recovery fund* ci dà l'opportunità di colmare ed è per questo che esorto i colleghi a votare la proposta di risoluzione che offre un *focus* molto dettagliato sul tema del mare e dell'economia blu, oltre che sulla biodiversità, e delle fondamentali azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

leggere tra le righe fumose ciò che vuole e chiaramente esprimere anche i propri desideri, ma poi bisogna affrontare la realtà.

Sappiamo che non basta soltanto parlare di *recovery:* servono soprattutto progetti e idee, ma non ne vediamo tante; ne vediamo soprattutto da parte degli italiani,

perché è un documento vecchio e superato, che non sarà presentato. Ecco perché noi di Fratelli d'Italia avremmo voluto un approccio completamente diverso e un pieno coinvolgimento del Parlamento, anche per presentare migliorie attraverso gli emendamenti.

un effetto totale sull'economia di circa 21 miliardi di euro. Bisogna lavorare - è fondamentale ed è uno dei temi che ho affrontato in Commissione ambiente e che continuo a sottolineare - soprattutto a una semplificazione dei vari procedimenti

Permettetemi di dire che hanno fatto sicuramente bene la Spagna, la Francia e anche il Portogallo: bisogna dare una prospettiva e un Governo deve avere anche lungimiranza nell'aiutare i nostri giovani. Questo non sarebbe un drammatico errore, ma una terribile occasione fallita, perché un Governo che non dà la possibilità ai giovani di rimanere in questo Paese di sicuro ha fallito completamente con le sue proposte.

Per l'espressione del parere in Commissione abbiamo contribuito notevolmente con i nostri suggerimenti, derivati anche dalle audizioni, a completamento di un lavoro già impostato dall'Esecutivo, che sicuramente sarà la conseguenza di tutti i progetti. I progetti previsti sono volti, in maniera preponderante, al rafforzamento della medicina territoriale - una scommessa e una sfida importanti e fondamentali - con la previsione delle case di comunità e il potenziamento dei servizi territoriali. Devono essere garantiti percorsi di prevenzione, diagnosi e cura per ogni persona, con un approccio basato sulla differenza di genere in tutte le fasi e gli ambienti della vita, quindi anche con un atteggiamento applicativo della medicina di genere. Ovviamente nelle case della salute e della comunità dovranno essere presenti professionisti competenti per materia, i quali dovranno riqualificare la loro formazione. Abbiamo detto tutti che la formazione è fondamentale e importante. Credo che il miglioramento del sistema sanitario

Credo che la sfida più importante sia però quella di calare sui territori in maniera concreta questi progetti, affinché possano davvero cambiare l'attuale situazione anche di disomogeneità. Mi riferisco a quanto stiamo vedendo anche con le vaccinazioni,

ripresa e resilienza sono note in libertà. Analizzo la situazione. Cari colleghi, qui in Italia abbiamo un buco potenziale che riguarda i derivati pari a 250 miliardi, di cui 181

che diventano tali dopo nove mesi di inesigibilità e per i quali la 6a Commissione, di cui faccio parte, ha giustamente auspicato un aumento dei termini (magari a diciotto

Può l'Europa emettere debito senza controllo del Parlamento tedesco? Questo ha bloccato tutto, per quanto riguarda la Germania. Si sa, vogliono comandare loro e infatti lo fanno. È una cosa grave questo comunicato, rispetto a quanto si dichiara. Come si finanzia l'Europa? Quando si sarà deciso di emettere questi 750 miliardi di titoli, andando a richiederli al mercato, l'Europa si finanzierà con l'intervento delle banche e delle istituzioni finanziarie internazionali, cioè con i nostri soldi finanzieremo noi stessi.

Non ho ancora capito bene - e mi farò violenza per il voto - la differenza tra prestiti e sussidi dei 209 miliardi. Non è ancora stata spiegata bene, o meglio lo è stata in qualche documento, ma facciamo finta di niente:

lavoro e passare alla transizione verde e digitale; queste sono cose auspicabili e condivisibili. Poi ci sono le priorità trasversali: la parità di genere, di cui sento parlare tanto in quest'Aula, i giovani e il

li daranno a *tranche*. Li avremo con qualche difficoltà, ma dobbiamo scegliere noi le opere. Ci sono degli elenchi. Scarseggiano le quote a favore degli enti locali. Ci sono 15 miliardi per la tutela del territorio e delle risorse idriche

il presidente Draghi sul famoso articolo del «Financial Times» per essere ottimista, un anno fa: bisogna fare insieme in Europa quello che si può fare, ma bisogna in primo luogo avere una strategia come Paese. Non bisogna lesinare l'aiuto alle famiglie e alle imprese, ma contemporaneamente occorre creare stimoli agli investimenti, perché solo questi ultimi possono creare posti di lavoro e quindi crescita e i posti di lavoro si creano anche con investimenti in settori non necessariamente generatori delle classiche fabbriche. Gli investimenti sulla sostenibilità sono ugualmente produttivi e creatori di posto di lavoro. Occorre attuare il vecchio che va bene e aprire al nuovo, con la semplificazione e la giustizia.

su 311 miliardi di risorse messe a disposizione dall'Unione europea per l'Italia. In particolare, dei 7,5 miliardi di euro che saranno erogati

«Agricoltura sostenibile», nell'ambito della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica». È evidente come oggi sia necessario lavorare affinché il ruolo dell'agricoltura venga riconosciuto come fondamentale e strategico,

Vediamo però di cosa stiamo parlando. Sono circa 750.000 le imprese agricole e i contadini coinvolti in questo progetto, che in Italia coltivano 12 milioni di ettari di terra. La dimensione media per azienda è meno di 15 ettari; ma ci confrontiamo con i vicini d'Oltralpe (la Francia), con 58 ettari per azienda, e con la Germania, dove ne abbiamo oltre 55. Questo è per dire che, quando scriviamo un documento, l'idea di difesa della produzione agricola italiana è diversa da quella di difesa dell'agricoltura europea, perché parliamo di dimensioni, di capacità produttiva e soprattutto di qualità e di sensibilità diverse. Poi sappiamo bene che la filiera del cibo in Italia vale quei famosi 540 miliardi, il 25 per cento del PIL, con un'importanza fondamentale. Il tema dell'inquinamento è trainante in questo documento e, da un punto di vista visionario, è a volte molto complicato. Anche su questo tema andiamo decisamente meglio, a livello di agricoltura, rispetto alla Francia e alla Germania. Gli agricoltori italiani emettono in atmosfera

aiutare i nostri agricoltori istituendo un fondo rotativo presso Ismea, al fine di sostenere l'accesso al credito delle aziende agricole per investimenti in innovazione e per gli stanziamenti mirati al rafforzamento delle politiche industriali di filiera,

per un valore di oltre 7 miliardi di euro. Ecco di cosa stiamo parlando; rischiamo infatti di fare un calderone di parole e di non riuscire a capire di cosa stiamo parlando. Nell'ambito della missione 2, abbiamo chiesto la promozione del biometano agricolo; è una sostenibilità e un'energia rinnovabile importantissima, attraverso la riconversione dei vecchi impianti. Abbiamo chiesto incentivi per il rinnovo delle macchine e dei mezzi circolanti, nonché alla riconversione irrigua e all'ammodernamento della rete. In certe Regioni solo l'1 per cento dell'acqua che cade dal cielo riesce a essere riutilizzata per l'irrigazione; non viene contenuta né trattenuta e nei mesi estivi ci sono grandissime difficoltà. Questa dev'essere una visione chiara per il futuro. Abbiamo chiesto il riconoscimento della strategicità delle filiere, con particolare riguardo alla zootecnia, al florovivaismo e alla filiera apistica, che è importantissima nel nostro Paese. Per il settore zootecnico devono essere messe in campo azioni volte ad aumentare la redditività delle singole imprese e degli allevatori. Abbiamo da poco audito l'Anaborapi in Commissione agricoltura (pochi minuti fa); si evince la difficoltà di un settore in cui non c'è il valore finale del prodotto che si produce e si lavora costantemente. È necessario avviare poi un processo di riforma della defiscalizzazione delle imprese che lavorano la filiera del legno. Nell'ambito della missione 3, abbiamo chieste alcune, comprese quelle portuali. Abbiamo chiesto la fine dell'isolamento di interi territori. Vengo da una provincia completamente isolata - la chiamano la terza isola d'Italia quella di Cuneo. Le infrastrutture sono fondamentali, come la logistica, anche e soprattutto per le imprese di trasformazione. Su questo tema, signor Presidente, vorrei dire che dobbiamo anche affrontare una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e una revisione della disciplina delle prestazioni occasionali, che semplifichi le procedure nell'utilizzo dello strumento. Guardando proprio alle sfide lanciate dall'agricoltura e dal piano del *green new deal*, è fondamentale considerare, al centro dell'importante processo di rinnovamento del settore, la figura dell'agricoltore, la sua costante presenza sul territorio, nel quale è fortemente radicato. Ciò rende questa figura importantissima per l'agricoltura, per l'ambiente e per il territorio, soprattutto perché ne è la prima e assoluta custode.

ricorderemo questi anni come i più duri della nostra storia recente. Questo terribile virus ha provocato nel mondo quasi tre milioni di morti, dei quali 107.000 sono nostri concittadini. Elevato è anche il tasso economico per le famiglie e le imprese, a causa delle pesanti conseguenze che ha portato con sé sull'occupazione, sul tessuto produttivo e sulla coesione economica e sociale. Sono state necessarie ingenti risorse per sostenere reddito e occupazione e rafforzare la sanità pubblica. Nel corso del 2020, sono state introdotte forme di sostegno che ammontano a 110 miliardi, corrispondenti al 6,6 per cento del PIL nazionale. Dinanzi a un evento di tale portata, però, questi numeri straordinari non bastano per arginare la crisi e favorire la ripresa. Abbiamo avuto bisogno di cooperazione sul piano di politiche economiche da parte dell'Unione europea. Siamo contenti di questa svolta, perché ha rappresentato un vero e proprio cambio di passo dell'Unione europea nel suo ruolo promotrice di politiche di coesione e di economia sociale. In questa prospettiva, il precedente Governo ha lavorato e ottenuto grandi risultati per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia da Covid-19, sappiamo che l'Italia sarà il primo beneficiario in termini di risorse per il piano straordinario Next generation EU e questo lo dobbiamo al grande lavoro che ha fatto il presidente Conte in Europa. Le ingenti risorse stanziate a questo fine sono un'occasione e, insieme, una responsabilità enorme. Non possiamo assolutamente sprecare l'opportunità di cambiare radicalmente questo Paese, a livello europeo, è stato il primo ad essere colpito, e anche più duramente. Siamo stati costretti a sacrifici personali, sociali ed economici per tutelare la salute pubblica ed evitare danni ancora peggiori. Le pesanti ripercussioni scaturite dalla pandemia hanno particolarmente colpito il settore del turismo e le attività ad esso collegate, azzerandone completamente i fatturati. Il Piano europeo per la ripresa e la resilienza mette in gioco una somma complessiva che ammonta a 225 miliardi; in sinergia con l'utilizzo di altre risorse europee, possono arrivare a oltre a 310 miliardi. Esaminando la proposta del PNRR in Commissione, circa gli aspetti prettamente competenti al turismo, emergono alcune debolezze che, nell'esame parlamentare, richiedono di essere compiutamente dettagliate e migliorate. Il nostro Paese è, senza alcun dubbio, una delle mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le sue condizioni climatiche, naturalistiche, socio-culturali, archeologiche, termali ed enogastronomiche. A fronte di queste potenzialità uniche, però, presenta in generale un'organizzazione turistica e soprattutto ricettiva non all'altezza di un tale patrimonio, quindi non in grado di produrre la ricchezza possibile. Se in tempi di prepandemia il fatturato

Gli interventi all'interno della componente 3 della missione 1 sono dedicati al tema del turismo e della cultura e prevedono l'utilizzo di complessivi 8 miliardi di euro. Aumentare nella totalità la quota degli investimenti destinati al rilancio delle imprese del turismo, potenziandone la concorrenzialità a livello internazionale, è prioritario. Di conseguenza, queste risorse devono essere utilizzate per colmare il *gap* digitale che, come in tutti i settori del nostro Paese, è ancora molto ampio, soprattutto in quelli del turismo e della cultura. Nell'ottica *green* e sostenibile delle nuove politiche varate a livello nazionale ed europeo, anche all'interno del patrimonio turistico ricettivo italiano, andrebbero estesi gli incentivi relativi alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica delle strutture del settore turistico. Ciò che si richiede è l'estensione della misura del superbonus del 110 per cento anche agli edifici che ospitano, per un miglioramento delle strutture turistico-ricettive

oltre a tenere conto delle potenzialità che può esprimere, prettamente turistiche, bisogna considerare anche ciò che rappresenta dal punto di vista sanitario. Il nostro Paese potrebbe vivere di turismo e di cultura. Un progetto minuzioso ed efficace di rilancio in questi settori rappresenterà un volano per l'intera economia italiana nell'era post-Covid-19. Per uscire da questa crisi e rendere l'Italia protagonista nella scena europea e mondiale, per il futuro delle nuove generazioni, occorre un progetto che sia innanzitutto coraggioso, chiaro e condiviso e che permetta al nostro Paese di ripartire e recuperare il terreno perduto durante il periodo della pandemia; occorre voltare pagina rispetto passato per avere un Paese moderno, all'avanguardia, verde, efficiente, sicuro ed ecosostenibile. Buon lavoro. credo che l'Aula semivuota sia la conferma dell'inutilità di questa seduta del Senato, che si trova a discutere di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che sicuramente non sarà quello che verrà presentato il prossimo 30 aprile a Bruxelles alle autorità europee. Già questo penso debba far riflettere i concittadini, gli italiani, di ogni linea politica e di ogni schieramento. Siamo qui a discutere di un PNRR che da mesi ci viene presentato come qualcosa di meraviglioso, un piano Marshall dei nostri tempi, del terzo millennio; un Piano nazionale di oltre 200 miliardi di euro (206, per la precisione). Vorrei ricordare però ai colleghi che hanno il piacere di ascoltarmi e ai cittadini che ci vorranno seguire che questo Parlamento ha già disposti in quest'ultimo anno

i risultati? Sono stati una totale assenza di risposte concrete sul tema dei trasporti, che tutti sappiamo quanto pesi sulla veicolazione del virus; virus; un'assenza di risposte sulla scuola, con i nostri figli, i nostri ragazzi ancora a casa in didattica a distanza; una campagna vaccinale

che hanno davvero immunizzato la propria popolazione, mentre noi siamo fermi, insieme agli altri Paesi europei, purtroppo ai soli nostri anziani (peraltro non a tutti). Non abbiamo dato risposte in termini di ristori prima e di sostegni ora, come diremo nei prossimi giorni. L'unica risposta che con i 180 miliardi abbiamo dato è stata in termini di *lockdown*,

ci troviamo a discutere di un PNRR che non è altro che quello trasmesso dal Governo Conte il 12 gennaio e che lo ha fatto cadere. Ebbene, oggi siamo qui di fatto a ragionare su un Piano nazionale di ripresa e resilienza che risponde a un Governo che è caduto proprio per effetto suo e a causa sua. Pensi che rispetto ha oggi il Parlamento.

Mi augurerei che almeno il Piano definitivo che verrà consegnato a Bruxelles innanzitutto venga in Parlamento. Lo ribadiamo noi di Fratelli d'Italia a voce alta: vogliamo che il Piano definitivo

il tema della digitalizzazione nel settore della riforma fiscale; i termini di interoperabilità delle banche dati; la piattaforma digitale per la cessione dei crediti d'imposta,

per incentivare l'arrivo della ricchezza e degli investimenti. Abbiamo avuto l'onore di vedere accolte le nostre proposte in materia di riforma fiscale nel parere della Commissione finanze. Speriamo che almeno nel PNRR definitivo, quello che verrà presentato in Europa, i temi della riforma fiscale abbiano adeguato riscontro.

la cosa più grave che possa accadere ad un'idea è che diventi un *brand*: succede quando certe idee spingono, perché impellenti al punto da non poter più essere ignorate; allora, vengono rubate proprio dai più ostinati detrattori, in una sorta di appropriazione indebita, per opposte finalità. È una strategia molto ben descritta ne «L'arte della guerra» di Sun Tzu: «quando il nemico cerca il vantaggio, getta l'esca per ingannarlo» e prosegue poi affermando che l'abile condottiero non segue uno schema prestabilito e non mantiene una forma immutabile, ma modifica la propria tattica adattandosi al nemico. Quando questo accade con l'ecologismo, si parla di *greenwashing*. Questo è esattamente il rischio che stiamo correndo oggi, che siamo giunti alla necessità, non più derogabile, di attuare una vera transizione ecologica, che ci transiti dal modello di sviluppo attuale, infinito in un mondo finito, ad uno circolare e in equilibrio, per superare e ribaltare il primo, che preme sul che preme sul pianeta con un'impronta ecologica insostenibile, che - come ci dicono gli studi - richiede le risorse di almeno due pianeti come il nostro e che ci porterà nel brevissimo tempo alla distruzione dei nostri stessi *habitat*. La crisi sanitaria è conseguenza del disequilibrio ambientale, perché un mondo malato non può che generare società malate e una società malata genera sistemi sociali ed economici malati e incapaci di dare risposte adeguate a tutti. Un disastro ambientale e socio-economico che colpisce già molti, ma che colpirà sempre più parti della popolazione mondiale: molte, moltissime persone, ma - ammettiamolo - non tutte. Moltissime terre verranno sommerse, altre invece si inaridiranno e dovranno essere abbandonate per il clima e la siccità; alcune forse geleranno, l'acqua sarà sempre meno e sempre più persone non vi avranno accesso. La capacità di alimentare diminuirà e sempre meno persone potranno essere sfamate. Le pandemie diventeranno strutturali ed endemiche e solo pochi Paesi industrializzati ad alto PIL potranno attrezzarsi per affrontarle e conviverci, con i vaccini che non sono per tutti. Non ci sarà più un posto per tutti sulla terra e c'è chi su questo dato sta costruendo un'ipotesi di società futura per pochi. Il rischio è che i fautori del modello produttivo attuale si travestano da paladini del cambiamento affinché nulla cambi e nessuno degli interessi finanziari globali che lo sostiene vengano davvero messi in discussione e intaccati, facendo anzi in modo di trarre da questo *brand* nuovi utili e futuri profitti. Il rischio è che il *greenwashing*, la mistificazione e la propaganda siano le armi spuntate con cui si proverà pericolosamente ad affrontare il cambiamento climatico. Dobbiamo prendere atto di questo: quella ai cambiamenti climatici e per l'ecologismo è una lotta di classe. Occorre che chi sta dall'altra parte della barricata si compatti, si unisca e giochi questa partita fino in fondo per vincerla. Per farlo è necessario tenere sempre presente che solo la giustizia ecologica ci potrà dare quella sociale e viceversa. Quella ecologica è una battaglia per i diritti, l'equità, la perequazione e l'inclusione. È la battaglia per un mondo più giusto per tutti. Infine, ma non per ultimo, signor Presidente, non possiamo tacere la necessità che questo processo dovrà essere guidato dal femminile che è dentro ognuno di noi. Il cambiamento di cui stiamo parlando dovrà essere sistemico e ciclico, olistico e inclusivo di tutte le parti e di tutte le relazioni. Non potrà essere un passaggio facile, governato solo da opportunità di mercato e da nuove filiere produttive, che pure saranno necessarie. Per passare però dal modello di sviluppo attuale, basato sulla competitività e sulla supremazia del più forte, a uno circolare e continuo, privo di scarti, basato sulla cooperazione, l'inclusione e la simbiosi, sarà necessaria una rivoluzione, prima di tutto culturale, non possiamo attuare senza riportare il femminile al centro del processo. Si badi bene: stiamo parlando di qualcosa di più delle pari opportunità o di un'equa presenza numerica di donne all'interno dei luoghi decisionali e di comando. Le donne sono naturalmente inclini al pensiero sistemico e resiliente, così come la nostra società dovrà imparare ad essere nel prossimo futuro. Il pensiero sistemico è lo specchio della nostra realtà, sempre più complessa e sempre più difficile da tenere in equilibrio, in una reciprocità di cause ed effetti, di perdite e di costi. È necessario adottare missioni di piano che valutino le azioni, le scelte e i progetti, in una relazione complessiva, sistemica e prospettica. *(Applausi)*.

tra le sei missioni del Piano, quella che ha un'attenzione particolare da parte dell'Unione europea, dunque anche per la trasposizione degli interventi nel nostro Paese, è proprio quella della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

tutto il campo delle energie rinnovabili e quindi l'abbattimento della CO2 e dei gas serra, superando il carbone, il petrolio e tutti i derivati.

il tema della mobilità sostenibile, anche locale, e quello della riqualificazione energetica e del recupero degli edifici. Nel nostro Paese, tre quarti degli edifici sono di classe energetica G, cioè la peggiore. Secondo stime fatte in maniera scientifica, ogni anno c'è un extra-costo di circa 20 miliardi di euro

i temi della rigenerazione urbana, della protezione del suolo e delle risorse idriche. Mentre stiamo parlando, nel 2021 ci troveremo nella situazione paradossale di non saper riqualificare le città e i centri urbani, che sono pieni di buchi neri, e contemporaneamente continuiamo a espandere la costruzione e il consumo di suolo vergine. Nel 2020 abbiamo consumato tanto suolo vergine quanto è estesa l'intera città di Bologna.

Certamente perché, grazie a dio, finalmente, a livello nazionale e internazionale, si è sviluppata l'idea che il nostro pianeta è una risorsa finita e che, di conseguenza, si pone il tema dello stato di emergenza ambientale e climatico. Proprio in quest'Aula, il 9 giugno dello scorso anno votammo la mozione sullo stato di emergenza,

e abbiamo migliaia di chilometri di coste. Per fare un esempio, a Venezia, la mia città, in questi cento anni il medio mare è più alto di 50 centimetri: 24 centimetri per la subsidenza, causata dall'emungimento delle falde acquifere, e 26 centimetri perché si alza il medio mare. Se uniamo questo ai fenomeni disastrosi legati al cambiamento climatico e quindi a quelli tropicali nel medio Mediterraneo e nell'Adriatico,

di Rio nel 1992 e con il Trattato di Parigi del 2015 e via dicendo, è diventata patrimonio comune. Non è solamente questo, però: l'Unione europea e il nostro Governo si sono resi conto che

perché la sostenibilità è amica dello sviluppo e del reddito. È questa la grande sfida culturale che dobbiamo portare avanti. Da ultimo, signor Presidente, mi soffermo sulla grande responsabilità nei confronti dei giovani: il PNRR, così come il *recovery fund*, è sulle loro spalle. Abbiamo la grandissima responsabilità di lavorare in modo tale che almeno gli investimenti che mettiamo a loro disposizione siano destinati a creare le condizioni per un futuro sostenibile e prospero, non solo per noi, ma anche per loro.

Signor Presidente, non le nascondo la mia difficoltà oggettiva a intervenire oggi, poiché arrivo da una terra, il cremonese, colpita nel cuore e negli affetti da questa pandemia. Proprio per questo motivo, il mio interesse per tale Piano è sempre stato alto e pieno di aspettative. Sento sulle spalle questa responsabilità quasi fosse una forma di rispetto per chi ha perso tutto: parenti, amici, lavoro. Oggi parliamo di quasi 200 miliardi è stato definito più volte dai *media* il nuovo piano Marshall del secolo. Proprio per questo, signor Presidente, voglio condividere con lei e con i senatori presenti in quest'Aula una mia semplice riflessione: 180 miliardi di scostamenti di bilancio bruciati in un anno, fatti a salti e singhiozzi di 30-40 miliardi alla volta; briciole da 600 euro ad alcuni e ad altri neanche quelli; categorie dimenticate, così come intere filiere, palestre, associazioni e piccole imprese. Potrei andare avanti e citarne migliaia, ma ecco il punto: 180 miliardi in un anno non li abbiamo neanche lontanamente considerati come una grande occasione, perché erano soldi nostri, mentre 198 miliardi in cinque anni li consideriamo il piano Marshall. Marshall. Credo che quei 180 miliardi fossero il nostro piano Marshall e mi permetto di dire una cosa al senatore che mi ha preceduto. Mi si permetterà di dire che una Nazione alquanto bizzarra non può non considerare questa cosa, così come - e non ha finito l'intervento, secondo me, dicendo che durante

di quei 180 miliardi di euro buttati all'italiana, vorrei che queste altre risorse fossero spese con criterio e in modo corretto; lo dobbiamo a tutti quelli che hanno sofferto e che stanno soffrendo per questa pandemia, che mi sembra non finire più. La politica, si sa, è l'arte di mediare e cambiare le cose, e lo fa sempre a modo suo; anche io faccio fatica a capire come ci riesca. Tuttavia, per la politica è sempre difficile cambiare le persone come me: è una sorta di odio-amore. Sono stato il primo a denunciare in Commissione lo scarso, se non nullo, coinvolgimento del Parlamento. Sono stato il primo ad alzare i toni sulla scarsa capacità del Parlamento di entrare nel merito del Piano. E ricordo ancora quei sorrisetti infastiditi degli ex Ministri alle mie parole e parlo non della preistoria, ma solo di qualche mese fa. Sono stato il primo a dire che il Piano doveva essere centrato non sul Mezzogiorno, ma sull'Italia intera, perché la pandemia ha colpito a morte iniziando la sua discesa proprio dalla mia terra e poi successivamente ha affamato tutto il Paese. Non dimentichiamolo mai questo. Non è più il momento delle divisioni: è il momento di far ripartire insieme il nostro Paese. Lei non sa e nemmeno immagina quanto mi sarebbe piaciuto essere qui oggi con un quadro di impegni e di investimenti chiaro, da votare con orgoglio, da far vedere alla Nazione. Quanto mi sarebbe piaciuto avere tra le mani un piano di investimenti che dicesse nero su bianco agli italiani, all'Italia intera, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quali sono i progetti, dove si sviluppano, quali per il Centro, quali per il Nord, quali per il Sud; quali saranno le ricadute economiche; quali saranno le analisi costi-benefici; come affronteremo le condizionalità. Oggi non abbiamo da presentare e da condividere tutto questo. Abbiamo audito quasi 300 persone, associazioni, Ministri, professori, comitati. Non ci siamo risparmiati su niente e di questo ringrazio il presidente Stefano, tutta la Commissione e le forze politiche che hanno partecipato, in un momento difficilissimo per tutti, fatto di zone rosse, di riunioni in presenza e a distanza. Io vorrei dare il mio contributo a questo Piano. È un mio dovere politico, civico e morale. Non voglio e non posso tirarmi indietro, perché non credo sia giusto. La politica deve responsabilizzarsi e alle volte fare scelte difficili. Oggi per me è una di quelle giornate fatte di scelte difficili: mi dovrò esprimere e dovrò indirizzare le mie decisioni sulla fiducia a un Piano di investimenti che, per un massimo di quasi 200 miliardi, verrà redatto da uffici tecnici; in sostanza, sarà quasi totalmente rifatto dai Ministeri; non sarà elaborato - come si vuol far credere - da questo Parlamento, che non lo ha nemmeno visto e non lo vedrà fino all'ultimo giorno utile prima di andare a Bruxelles per essere presentato, ma che responsabilmente se ne sta prendendo di fatto la paternità. Mi farebbe male, signor Presidente, scoprire un giorno che i nostri figli siano messi in condizione di pagare la scelta strategica che ha fatto un tecnico, perché quel benedetto tempo di lavorare in modo diverso purtroppo non c'era e non c'è mai. Capisco, dall'altra parte, le difficoltà del nuovo Governo ad affrontare in trenta giorni un lavoro che, come minimo, doveva durare otto Capisco e vedo un lavoro, il precedente *recovery plan,* totalmente sbagliato, partito sul nascere in modo sbagliato, sottovalutato e lasciato inevitabilmente in mano a burocrati che stanno cercando di riscriverlo. Io sono moralmente costretto a votare la proposta di risoluzione di maggioranza proprio per il discorso di responsabilità che ho fatto prima, ma non posso permettere che il Paese perda anche un solo centesimo di quel Piano di investimenti. Spero solo che quegli uffici abbiano lavorato e lavorino in questi ultimi trenta giorni con la stessa tenacia e volontà che ci ho messo io e ci ha messo la Commissione. Abbiamo consegnato 73 pagine di relazione congiunta, più allegati e dettagliate relazioni delle Commissioni. Si tratta di una mole di lavoro gigantesca; auspico e tenga conto delle segnalazioni che abbiamo fatto pervenire. Avviandomi alla conclusione, come diceva sant'Agostino, signor Presidente, la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio: lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle

vorrei portare all'attenzione di quest'Assemblea alcuni aspetti nell'ambito del tema della sanità. Abbiamo parlato di potenziamento della rete ospedaliera.

La pandemia, oltre ad aver evidenziato le gravi criticità della nostra medicina territoriale, ha anche letteralmente travolto - e sta continuando a farlo già negli anni precedenti, ogni inverno - lo dico anche per esperienza, e c'è la testimonianza dei nostri colleghi - gli ospedali erano travolti dalle epidemie influenzali: influenzali: non si trovava più un posto letto e, quindi, si avevano lunghe attese ai pronto soccorso, malati in barella, nei corridoi, negli atri, in ogni spazio disponibile.

le terapie intensive, ma anche le degenze ordinarie e le semi-intensive, che hanno un certo grado di flessibilità e sono molto poco rappresentate in Italia, ma per far fronte a eventuali pandemie possono essere molto importanti.

L'epidemia Covid ha reso necessarie nuove assunzioni: circa 37.000. Tuttavia, questo personale rimane tuttora in gran parte precario. Quindi, se vogliamo garantire continuità, sicurezza, qualità delle cure dobbiamo fare in modo che questo personale faccia parte stabilmente degli organici.

non trovano poi attrattivo e soddisfacente il lavoro nel nostro Servizio sanitario nazionale, per cui si rivolgono al privato e molto spesso all'estero.

Un ultimo aspetto molto importante concerne le liste d'attesa. Sappiamo tutti che nell'era Covid, purtroppo, molte prestazioni (*screening* come visite ambulatoriali,

- interventi alla prostata - non per casi oncologici - per cui le persone aspettano mesi, anche anni, con i disagi e i rischi di complicanze dovute al fatto di dover portare un catetere vescicale a permanenza. questo caso è necessario un intervento, una pianificazione in modo da ripristinare l'accessibilità alle cure. Quindi, ben venga la medicina territoriale e il suo potenziamento. Ben venga la sanità di prossimità,

se l'Italia non risolve i gravi problemi della giustizia, sarà molto difficile garantire una vera ripresa economica. Sappiamo tutti molto bene che gli investimenti, soprattutto quelli che provengono dall'estero, sono legati all'efficienza e alla rapidità con cui il nostro sistema giudiziario sarà in grado di dare risposte alla domanda di giustizia. Purtroppo, oggi, non è così,

di risorse per la giustizia ce ne sono troppo poche. È vergognoso che per la giustizia si preveda appena l'1 per cento o poco più dell'intero *recovery fund*.

onoraria. Abbiamo 5.000 professionisti altamente specializzati, formati in anni e anni di lavoro sul campo, che stiamo trattando come fossero i *rider* della giustizia, ossia senza diritti,

la riforma del Consiglio superiore della magistratura. A causa delle vergognose vicende che tutti conosciamo hanno perso fiducia nella giustizia. Bisogna porre fine alla lottizzazione correntizia e al mercimonio delle più alte cariche della magistratura, provvedendo a una riforma radicale

politica e magistratura, tra magistratura e politica. Il magistrato che si candida alle elezioni politiche o amministrative - che venga eletto o meno - avendo fatto una scelta di parte non può tornare a svolgere funzioni giurisdizionali, deve essere collocato fuori ruolo nei Ministeri, negli organi costituzionali e nelle ambasciate. Non può tornare a rendere giustizia nei tribunali, né svolgere funzioni requirenti perché i cittadini hanno diritto di avere fiducia nella giustizia e nell'imparzialità di chi li giudica. giudica. Infine, bisogna mettere mano alla legge che limita in modo vergognoso la responsabilità civile dei magistrati. Anche i magistrati, se sbagliano, devono pagare.

Fratelli d'Italia, da opposizione responsabile e patriottica, è disposta a collaborare nell'interesse superiore della magistratura. Se invece non avrete questo coraggio, noi saremo sempre qui a denunciarlo e incalzarvi. *(Applausi)*.

Il rapido susseguirsi di due crisi finanziarie e di un'emergenza sanitaria di proporzioni globali ha avuto pesanti conseguenze sull'occupazione, sul tessuto produttivo, sulla coesione economica e sociale di tutti i Paesi nel mondo. In questo anno e mezzo abbiamo potenziato le capacità di risposta del Sistema sanitario. Abbiamo imparato come modulare le restrizioni per fronteggiare il virus. Siamo più strutturati nell'affrontare l'emergenza. Oggi, però, con questo atto siamo chiamati a chiarire quale deve essere la prospettiva. Mi riconosco nelle parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: si tratta non solo di riparare e recuperare l'esistente, ma anche di plasmare un modo migliore di vivere nel mondo di domani. Il compito storico a cui siamo chiamati è costruire l'Unione europea e l'Italia per le prossime generazioni. Per l'Italia in particolare si tratta di voltare pagina rispetto al passato. Oggi indichiamo in maniera chiara che non ci possiamo limitare alla ripresa post-Covid, porre le basi dell'Italia del futuro, l'Italia dei nostri figli, dei nostri nipoti e pronipoti. Nell'ottica del concetto dello sviluppo sostenibile, dobbiamo salvaguardare quanto è stato costruito fino ad ora e valorizzare le tantissime risorse che finora non sono state utilizzate in pieno. Penso al Mezzogiorno d'Italia e alle Regioni con tassi di sviluppo inferiori a quelli nazionali. Occorre creare posti di lavoro stabili, con investimenti strutturali in progetti di sviluppo sostenibile che guardino al futuro. Non abbiamo bisogno di tanta fantasia per individuarli: basta valorizzare risorse primarie quali i prodotti agricoli, le bellezze naturali, il grande patrimonio culturale frutto di millenni di storia e tradizioni. Tra l'altro, queste risorse hanno la caratteristica che non possono essere delocalizzate e quindi sono disponibili per attrarre investimenti stranieri che in Italia stentano ad arrivare, principalmente a causa della complessità del nostro sistema burocratico e per la mancanza di certezza del diritto: questioni che oggi vanno affrontate con coraggio e determinazione. Mi permetto ora, Presidente, di parlare di una delle più grandi risorse dell'Italia: il turismo. L'Italia è senza dubbio la destinazione preferita in tutto il mondo. Io che vivo all'estero posso affermare che c'è grande fame di Italia nel mondo e, quando le restrizioni ai viaggi internazionali saranno rimosse, ci sarà una grande massa di persone che ha tanta voglia di viaggiare e visitare anche il nostro Paese. Penso quindi che dobbiamo porci tre obiettivi: il primo è salvaguardare la rete di strutture del settore che ha permesso all'Italia di essere uno dei Paesi più visitati al mondo; dobbiamo aiutare le strutture ricettive, gli operatori turistici e gli enti culturali che oggi sono fra le categorie più colpite dalla crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia. Il secondo obiettivo è intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero e incoraggiarli a estendere la loro visita dell'Italia a luoghi bellissimi e interessanti che fino ad oggi non hanno fatto parte dei tradizionali itinerari turistici. Mi riferisco ai tantissimi borghi, boschi, spiagge, siti archeologici che rendono il nostro Paese unico al mondo. Occorre orientare i visitatori verso le piccole e medie città d'arte e verso itinerari turistici regionali. Il terzo obiettivo è la promozione dell'Italia nel mondo. In generale, l'Italia si promuove da sé, non abbiamo bisogno di tanta fantasia. Abbiamo invece necessità di far conoscere i piccoli centri anche dell'entroterra, le tipicità, gli usi e i costumi tipici dei luoghi, le manifestazioni culturali proprie di quei posti. Rispetto alle altre Nazioni abbiamo un grande vantaggio: 70 milioni di cittadini italiani e discendenti di cittadini italiani vivono nel mondo. Si tratta di una grande risorsa che dobbiamo valorizzare. Sono i nostri ambasciatori nel mondo, fortemente legati alle loro origini. Non perdono occasione per promuovere il nostro bellissimo Paese nelle comunità in cui vivono. Loro stessi rappresentano una grande risorsa di turismo: il cosiddetto turismo di ritorno. C'è tanta voglia dei nostri figli e nipoti di venire in Italia a riscoprire i luoghi di origine dei loro genitori e nonni. Io penso quindi che dobbiamo puntare su una campagna di promozione all'estero seguendo due direzioni: da un lato, mirare alla diffusione di informazioni attraverso la stampa e i media locali, editi anche in lingua italiana; alla produzione di materiali specifici per turisti che hanno voglia di scoprire nuovi luoghi; alla promozione del territorio attraverso le tantissime agenzie di viaggio specifiche, molto spesso gestite da nostri connazionali. Dall'altro lato, occorre investire in lingua e in cultura: investimento e non spesa. Occorre promuovere l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole locali a tutti i livelli, dalle scuole primarie all'università; produrre materiale didattico e informativo che possa essere utilizzato nei corsi di lingua; promuovere iniziative di turismo sociale, gli scambi culturali tra scuola e università; promuovere iniziative culturali in grado di produrre un impatto nelle società locali e rimuovere gli ostacoli all'accesso dei programmi televisivi italiani in *streaming*. In questo investimento dobbiamo coinvolgere tutto il *network* degli italiani all'estero, costituito dalla rete delle camere di commercio, dalle istituzioni di rappresentanza, dai *media* in lingua italiana, dagli operatori turistici. Nello stesso tempo, però, dobbiamo investire in Italia, innanzitutto per migliorare la viabilità interna e locale, che aiuta a raggiungere borghi e piccoli centri che possono sembrare a volte isolati. Occorre costruire nuove strutture ricettive, promuovendo la nascita del cosiddetto albergo diffuso ed ecologico anche nei centri storici, che potrebbero avvantaggiarsi dei finanziamenti dell'ecobonus. Tutto ciò è possibile se si uniscono le energie e gli investimenti degli enti territoriali e nazionali (Stato, Regioni ed enti locali). I nostri concittadini nel mondo, oggi come nel passato, potranno contribuire alla nostra economia con risorse economiche dall'estero: rendiamoli protagonisti di questa nuova rinascita del Paese. Signor Presidente, membri del Governo, gentili colleghe e colleghi, innanzitutto un ringraziamento ai Presidenti e ai membri delle Commissioni 5a e 14a, che hanno dovuto elaborare in così breve tempo le osservazioni pervenute dalle altre dodici Commissioni; il lavoro di analisi e di sintesi finale di tutte le osservazioni sarà stato di non poco momento. Rivolgo un ringraziamento anche ai funzionari, che spesso dimentichiamo di ringraziare per il loro contributo determinante. Ho davanti a me tre documenti su cui mi piacerebbe spendere i prossimi minuti del mio intervento, che hanno al centro l'interesse verso la questione della della transizione energetica, e più precisamente l'analisi dell'indirizzo politico che noi comunicheremo attraverso le risoluzioni che approveremo

e le ultime dichiarazioni del ministro Cingolani, che ieri, in occasione di un evento digitale organizzato da «Il Sole 24 Ore», ha esternato i propri pensieri e le proprie considerazioni sulla tematica in oggetto. Devo innanzitutto dire che il contenuto della relazione

nel senso che si osserva un'attenzione alla tematica e una volontà di identificare gli obiettivi da raggiungere, come - ad esempio - ridurre la dipendenza

fini sperimentali, in attesa del recepimento della direttiva comunitaria RED II. Ora, se è vero che nei prossimi mesi probabilmente recepiremo completamente la direttiva sulle fonti rinnovabili, è anche vero che fortunatamente il nostro Parlamento ha già adottato misure normative volte all'introduzione della operatività già attuale delle comunità dell'energia e dell'autoconsumo collettivo. Sono normative purtroppo ancora misconosciute, anche da parte dei tecnici, perché approvate nel corso del periodo pandemico e che hanno bisogno di ulteriore approfondimento. Queste possibilità, che già esistono nel nostro ordinamento, vanno giustamente potenziate e valorizzate, come indica la relazione. Così come mi piace vedere che si invita il Governo a sostenere lo sviluppo dell'idrogeno verde, cioè quello prodotto da fonti rinnovabili, in un'ottica realistica dove l'idrogeno prodotto dal metano (il cosiddetto idrogeno blu), che non può ovviamente essere vietato e che sappiamo bene essere oggi il 95 per

il Parlamento qui ribadisce, è che gli impegni finanziari relativi al potenziamento dell'idrogeno verde vedono le somme indirizzate solo per lo sviluppo di quella fonte energetica, e cioè dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. In quelle schede tecniche mi piace vedere che si indica anche un obiettivo di potenza installata da elettrolizzatori,

ambizioso possa rimanere nella disponibilità di società straniere, perché sarebbe veramente un peccato. C'è un obiettivo, al 2030, di 5 gigawatt di potenza installata,

da impiegare per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Quello che forse manca è un obiettivo intermedio, quello che l'Europa identifica, nel 2024, come 6 gigawatt. Sarebbe bene che l'Italia identificasse anche quell'obiettivo intermedio. Infine, il ministro Cingolani si muove indubbiamente su questa linea nel momento in cui riconosce che l'idrogeno è un treno internazionale dal quale non possiamo chiamarci fuori, in prospettiva, come come vettore di energia assolutamente pulito. Quindi, il finale di questa storia - come anche il Ministro stesso ci ricorda e come pure nella relazione è indicato - è che occorrerà, per poter correre, veramente un'azione decisa su semplificazione e permessi, e cioè incidere a livello normativo e regolamentare

occorrerà produrre molta più energia elettrica da impianti eolici - sono previsti anche quelli *off-shore* - e da impianti fotovoltaici, con le *hydrogen valley* previste nella versione attuale del PNRR, per poter raggiungere quegli obiettivi ambiziosi a cui dobbiamo tendere tutti. Al momento, ripeto che continueremo a vigilare e a coordinarci con il Governo affinché questi obiettivi siano rispettati e, se possibile, anche migliorati.

Per la Lega è importante che, oltre all'obiettivo principale della neutralità climatica, si punti a come ridurre la dipendenza energetica del Paese troppo alta; a come ridurre il costo delle bollette, le più alte in Europa; a come ridurre l'inquinamento dell'area del bacino padano; a come tutelare le nostre filiere nazionali. Il Piano, che il Governo Conte ci ha lasciato pieno di lacune, deve essere rivisto anche per essere coerente con il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), che deve essere anch'esso aggiornato con *target* più sfidanti rispetto ai vigenti, che, peraltro, abbiamo già difficoltà a raggiungere. Sulle rinnovabili, in Italia lo sviluppo non va bene. I dati pubblicati ieri registrano, nel 2020, un calo delle installazioni del 35 per cento rispetto al 2019: e non è solo colpa del Covid-19. Da qui al 2030 dovremmo installare ogni anno nuovi 5 gigawatt. Invece, andiamo a una velocità da lumache inferiore del 20 per cento a quanto dovremmo. Le aste DM FER1 per gli incentivi sono un fallimento e il confronto con la Spagna è impietoso. Se aspettiamo le rinnovabili, di questo passo altro che idrogeno verde: non riusciremo nemmeno a spegnere le centrali a carbone al 2025. Occorre, soprattutto, rimuovere gli ostacoli per chi vuole investire, semplificando gli *iter* autorizzativi, intervenendo anche sui procedimenti di VIA e sull'azione di interdizione operata dalle sovrintendenze. Sull'idrogeno, in tanti sostengono che l'Italia sia pronta a questa sfida. Io ho tante perplessità. Ci sono forze politiche, a partire dai 5 Stelle, che vogliono solo quello verde, ma questo avrà un ruolo importante solo nel lungo termine. Che piaccia o no, sarà il gas a esercitare il ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. È dunque stucchevole la contrapposizione in atto su quale idrogeno sostenere a breve (verde, blu, rosa o grigio). Se vi è consapevolezza che l'idrogeno è importante per la decarbonizzazione, allora, in attesa che maturi la tecnologia, è sbagliato assumere una scelta unidirezionale. Oggi infatti l'idrogeno verde non è competitivo. Hai voglia a parlare di idrogeno per il rilancio dell'Ilva: ne risulterebbe un aumento spropositato del costo dell'acciaio, devastante dal punto di vista competitivo rispetto a quello turco-cinese. Manca ancora una strategia italiana su questo vettore energetico: non si è ancora deciso dove produrlo, come trasportarlo, da parte di chi e come utilizzarlo, visto che non c'è ancora un mercato. Inoltre, per idrogeno verde c'è carenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: non abbiamo i kilowattora verdi per gli obiettivi del PNIEC, figuriamoci per l'idrogeno. L'Italia non ha l'eolico della Germania e il nucleare della Francia. Per l'efficientamento energetico c'è ancora tanto da fare e, sul superbonus, al momento di super esistono solo i problemi, i superproblemi, creati da una misura tanto sbandierata quanto complicata, che non sta dando quello *shock* atteso dal settore edilizio. È assolutamente necessaria una proroga, almeno al 2023, diversamente non parte più nessuno, figuriamoci i condomini. Serve assolutamente una semplificazione, almeno per risolvere il problema delle difformità edilizie. Per la mobilità sostenibile non possiamo pensare solo all'elettrico, che - lo sottolineo - inquina anch'esso nel suo ciclo di vita, a partire dalle batterie, oggi per il 70 per Non solo stiamo affossando la nostra filiera dell'*automotive*, già in crisi per il Covid-19, ma il corposo sostegno all'acquisto di un'auto elettrica, bene di lusso, con *bonus* che vanno oltre i 10.000 euro, rischia fortemente di aumentare le disuguaglianze sociali. Alla fine del 2020, a forza di incentivi, abbiamo messo in strada poco più di 70.000 auto elettriche. Ma voi pensate veramente che sia sostenibile, come scritto nel PNIEC, raggiungere al 2030 i quattro milioni di auto elettriche, oltre ai due milioni di ibride *plug-in*? Dove troviamo i 60 miliardi di euro di soldi pubblici? Allora, per decarbonizzare il settore dei trasporti, in attesa dell'idrogeno, è doveroso - e lo dice anche il PNIEC - sostenere lo sviluppo dei biocarburanti e dei carburanti sintetici, l'uso del GPL, del gas, del biometano, che proprio l'altro ieri la Commissione europea ha incluso quali combustibili per alimentare le auto pulite che possono beneficiare di incentivo, oltre ai diesel di ultima generazione. Dunque, altro che bando dei veicoli a combustione interna, a maggior ragione se a bassa emissione. Una domanda per chi pensa sempre in *green*. Il parco circolante italiano al 2020 conta 40 milioni di auto; di queste, 30 milioni sono vecchie, tra euro 0 e Interessa a qualcuno il loro inquinamento, a parte bizzarre proposte di imporre il divieto di circolazione? Stiamo scherzando con la crisi che c'è? Milioni di proprietari non hanno soldi per acquistare un'auto nuova, figuriamoci una elettrica. Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con tre brevi riflessioni. Mettiamo in campo tutto il pragmatismo e lasciamo perdere costose derive ideologiste, inefficaci e anti-impresa; diversamente falliremmo con il Piano e sprecheremmo tanti miliardi. Occorre che il Governo, nella redazione finale del Piano, consideri le indicazioni contenute in questa equilibrata relazione, di cui alcune molto importanti della Lega, e coinvolga il Parlamento per il monitoraggio degli stati di avanzamento, degli impatti e delle analisi costi-benefici. Sappiamo, poi, che il Governo sta lavorando a un nuovo decreto semplificazioni: attenzione a non fare un *omnibus*. Non possiamo pensare in questa fase di dare una sferzata a tutti i mali della burocrazia, perché rischieremmo di fare un buco nell'acqua. Puntiamo dunque a riforme mirate. Terza e ultima riflessione: l'Europa sia prudente nel voler fare sempre la prima della classe. È responsabile solo del 10 per cento delle emissioni di CO2 e le *policy* troppo spinte alla decarbonizzazione rischiano di mettere ulteriormente in ginocchio le nostre imprese. Al contrario la Cina, che con il 30 per cento di CO2 è il più grande inquinatore del pianeta e continuerà ad esserlo, mentre noi spegniamo le centrali a carbone, ne costruisce di nuove. *(Applausi)*. Lo scorso anno ne sono spuntate cinquanta e in progetto ne hanno ancora una sessantina. A loro interessa produrre a bassi costi. Non lamentiamoci dunque se Pechino acquisterà nel commercio globale sempre più quote di mercato e si rafforzerà, lavorando per spostare

Signor Presidente, signora sottosegretario Sartore, colleghe e colleghi, la stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci ha posto di fronte l'importante compito di rivedere l'assetto del Servizio sanitario nazionale in prospettiva di una più adeguata corrispondenza alle sfide che minacciano la nostra salute; temi trattati nella missione sei «Salute» del Piano, nella cui componente C1 sono previsti interventi di potenziamento dei modelli di assistenza alle cure primarie. È positivo e giusto che l'assistenza socio-sanitaria possa svolgersi, laddove possibile, prioritariamente a casa del malato ed è doveroso creare le condizioni perché ciò avvenga omogeneamente in tutto il territorio nazionale, costituendo un valido sistema di assistenza in rete, in grado di rispondere ai bisogni di persone fragili e di pazienti cronici, trattabili a domicilio attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, supportata dall'impiego di modelli digitali per soluzioni di telemedicina e *connected care,* fondamentali per il monitoraggio e la diagnosi a distanza dei pazienti. È giusto quindi che le risorse del *recovery fund* vengano impiegate per garantire e potenziare le prestazioni domiciliari H24, per trecentosessantacinque In questo modello di assistenza territoriale le case di comunità e gli ospedali di comunità costituiranno altri presìdi fondamentali nei quali verrà data risposta alle esigenze di salute di pazienti che non abbisognano di cure complesse come quelle ospedaliere, ma che comunque necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria; strutture pertanto dotate di posti letto per malati cronici non autosufficienti, per malati dimessi dagli ospedali che non possono rientrare al domicilio, per esigenze di riabilitazione e-o lungodegenza, o ancora nuclei residenziali per cure palliative e ricoveri di sollievo, per una completa presa in carico dei malati affetti da malattia in stadio avanzato. Poiché la salute degli uomini non può essere disgiunta dalla salute e dalla qualità dell'ambiente, anche il nostro ambiente di vita dovrà migliorare, in particolare le città, divenute negli ultimi decenni fonti di squilibri sociali e di grave inquinamento. Esse devono essere reinterpretate in termini di rigenerazione urbana. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con gli obiettivi europei e dell'Agenda ONU 2030, prevede anche interventi per rendere gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri e sostenibili a consumo di suolo zero. Un altro aspetto della componente territoriale C1 della missione «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anch'esso fondamentale per migliorare la nostra qualità di vita, consiste nell'approccio *one health*, che affronta in visione unitaria le correlazioni tra salute e ambiente, benessere e clima. È apprezzabile l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute, ambiente e clima (Snpsa), con i conseguenti atti applicativi e attuativi che consentiranno, attraverso l'attuazione con l'attuale Sistema nazionale protezione ambientale, di gestire la tematica salute e qualità dell'ambiente, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese. In questo contesto si auspica che venga data immediata attuazione alla costituzione, all'interno dei dipartimenti di prevenzione di tutte le aziende sanitarie nazionali, di unità operative di medicina ambientale, costituite da medici e tecnici specialisti in grado di affrontare adeguatamente questioni di salute correlate agli ambienti di vita. Si ritiene non ulteriormente procrastinabile promuovere la formazione medica specifica mediante il finanziamento di otto borse di studio di specializzazione post-universitaria in tema di medicina ambientale confidando nella loro implementazione nel tempo. La conoscenza dei nostri ambienti di vita, la prevenzione sanitaria e l'educazione ambientale devono essere pilastri della ricostruzione dello stato sociale. Bisogna pensare in termini concreti alla relazione tra la salute e l'ambiente e al mondo che stiamo lasciando alle nostre generazioni future e considerare che tutto quello che si investe oggi in prevenzione sarà non soltanto un guadagno di salute domani, ma anche un risparmio di finanze per tutti i capitoli di bilancio dello Stato. Al fine di dare concreta attuazione e forza a questi progetti, riteniamo anche necessario e prioritario riportare la *governance* della salute nell'alveo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ricordando peraltro che in materia di profilassi internazionale l'assetto delle competenze, fin dagli articoli 6 e 7 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *q)*, della Costituzione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono dinanzi a una malattia pandemica. Non è più giustificabile mantenere disomogeneità e squilibri di comportamento delle varie Regioni e Province autonome, come quelli ai quali si è dovuto assistere in questi ultimi mesi, perché comportano gravi compromissioni di diritti fondamentali di tutti i cittadini, ancora più gravi se si ripercuotono sulle categorie più fragili e indifese. Inoltre, il ritorno alla centralità dello Stato di tutte le attività sanitarie sicuramente eviterebbe il ripetersi di spiacevoli e gravi avvenimenti, come quelli accaduti nei giorni scorsi nella Regione Sicilia, in merito ai quali ci auguriamo che la magistratura faccia piena luce, individuando colpe e responsabilità. *(Applausi)*.

È un Piano ambizioso, con in teoria grandi mezzi, che non può trascurare alcuna questione. Forza Italia, nel consegnare le sue proposte al Presidente del Consiglio, ha evidenziato la necessità di individuare anche risorse adeguate. Della Capitale si parla poco nei documenti che circolano; viene soltanto evocato a un certo punto il ruolo di Roma *caput mundi* - si usa questo termine per la tutela del patrimonio artistico e culturale. Certamente Roma da questo punto di vista rappresenta uno dei tesori del pianeta e quindi è giusto menzionare il patrimonio artistico e culturale della Capitale d'Italia. Ma - a nostro avviso - è necessario anche cogliere l'occasione per dare finalmente alla Capitale un ruolo definito, perché c'è bisogno di rilanciarne la funzione. C'è un debito pesantissimo che accompagna la vita di questa città e pesa anche la mancata attribuzione di poteri specifici che ogni capitale europea ha in quanto capitale dello Stato. È un'antica questione: Roma, per le responsabilità che ha, perché ospita Ministeri, ambasciate, sedi internazionali e ha oneri di ogni genere, non può essere gestita,

ci fu un'ultima occasione nel 2019 con un emendamento al decreto crescita che fu respinto dalla maggioranza dell'epoca - ma insistiamo perché si assegnino poteri diversi alla Capitale. Il Governo Berlusconi con una legge del 2009 intervenne in tal senso, ma in questa legislatura, come in altre precedenti, è stato presentato un disegno di legge costituzionale per modificare l'articolo 114 della Costituzione e dare a Roma poteri simili a quelli di una Regione. Su questo Forza Italia insiste, perché un assetto diverso è utile alla Nazione. ospita e ospiterà, quando il mondo riprenderà la sua vita normale, eventi di ogni rilievo e di ogni natura. È anche la Capitale della cristianità, oltre a tutto il resto. Nel 2025, che in termini organizzativi è domani mattina, ci sarà un Giubileo, che potrà essere anche importante per rilanciare la funzione della Capitale e dell'Italia, anche per la sua rilevanza morale. Roma ha bisogno di infrastrutture e di una mobilità sostenibile. L'elenco delle opere che abbiamo indicato nella nostra proposta di *recovery plan* è molto lungo: dall'anello ferroviario al finanziamento della metro D, alla metro A, alla metro B e a un nuovo progetto di linea E. Roma è in ritardo rispetto ad altre capitali internazionali come rete di metropolitana. Anche le metrotranvie di superficie devono essere assolutamente potenziate. C'è il tema poi della rigenerazione urbana, che si sta discutendo al Senato con un disegno di legge assurdo, che oggi è attualmente in discussione presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che va riscritto. La rigenerazione urbana vuol dire ristrutturare edifici, ricostruirli, salvaguardando ovviamente le parti di pregio artistico e storico dei centri cittadini. A Roma, con un emendamento nel decreto semplificazione del Governo giallorosso, si è paralizzata la zona A, che non è solo il centro storico in senso stretto, che ha un valore storico, culturale e architettonico di pregio, ma è praticamente tutta la città, impedendo ristrutturazioni e rigenerazioni, che sono - quelle sì - la transizione ecologica e non quella demagogica che viene evocata. *(Applausi)*. Ciò vuol dire risparmio energetico, riscaldamenti che possono essere gestiti diversamente e cappotti termici. La rigenerazione urbana è un tema nazionale e internazionale molto sentito il Governo Conte ha paralizzato la Capitale. Anche il PD ha votato, insieme ad altri, l'articolo 10 del decreto semplificazioni, che è distruttivo, antiecologico e demagogico. Non si può inneggiare alla transizione ecologica e digitale e opporsi alle politiche di

debba entrare nel *recovery plan*. Abbiamo posto questo tema anche al Presidente del Consiglio, che certamente è uomo europeo per eccellenza, anche per la sua opera degli ultimi anni, apprezzata da tanti, ed è anche un romano. È ovvio che questo non è un discorso campanilistico: se Roma è la Capitale, deve avere una dotazione normativa e di mezzi che ne giustifichi il ruolo e la proietti nell'interesse della Nazione intera. Presidente, concludendo, ho voluto dedicare il mio intervento a questo tema, augurandoci che nel Piano possa avere una maggiore forza. Lo abbiamo chiesto al presidente Draghi e lo chiediamo in questa circolazione

poco tempo a disposizione, cercherò di utilizzarlo quantomeno per rimettere al centro ciò che riteniamo sia molto importante, almeno per il nostro partito, e cioè la questione delle infrastrutture. In questi giorni tutti abbiamo avuto modo di di assistere al disastro economico causato dal blocco del Canale di Suez. Abbiamo visto una fotografia devastante, perdite miliardarie, che ci fanno ripensare a una economia reale, vera e concreta, fondata sul lavoro, sull'ingegno e sul sacrificio umano, così diversa da quella figlia dell'alta finanza e dell'interesse sul debito, che, purtroppo, troppo spesso incide sulle nostre esistenze. Ripartirei da quel quadro, dall'importanza delle infrastrutture, soprattutto per una Nazione, come quella italiana, che ha una posizione del tutto privilegiata,

tantissimo spazio da questo punto di vista. Le navi oggi attraccano e partono in altri porti, nonostante l'Italia sia una piattaforma ideale al centro del Mediterraneo. Stiamo perdendo, secondo gli ultimi dati, qualcosa come 70 miliardi di euro all'anno per carenze infrastrutturali.

collegare la nostra Nazione e soprattutto di dare la possibilità al genio italiano, ai nostri lavoratori e ai nostri imprenditori di cimentarsi in imprese che solo noi possiamo A Genova abbiamo dimostrato come gli italiani sanno reagire, costruendo un ponte in pochissimo tempo. Adesso credo che siamo pronti per il ponte sullo Stretto, altra battaglia di Fratelli d'Italia e dei patrioti che sicuramente può ridare lustro e rilancio alla nostra Nazione. Credo che dobbiamo interrogarci su questo e metterci alla prova. Ci sono tanti soldi, la stragrande maggioranza dei quali dobbiamo restituire, quindi investiamoli bene.

oggi stiamo discutendo del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, un progetto presentato il 15 gennaio 2021,

abbastanza grave, poiché presenta ancora numerose lacune e certamente la Commissione europea non potrebbe accoglierlo favorevolmente. Se questo Piano, per come oggi è strutturato, venisse presentato alla Commissione europea così com'è sicuramente verrebbe respinto con diverse osservazioni. Purtroppo questo non farà altro che aggravare la situazione dell'Italia, che ha già serie difficoltà nella spesa dei fondi europei che ogni sette anni vengono assegnati ai vari Paesi membri. Mi riferisco ai fondi del 2014-2020: l'Italia ha speso solamente il 38

invece di poter spendere adeguatamente investendo in sviluppo e crescita per il nostro Paese ben 191 miliardi?

sono a prestito mentre 68,9 miliardi saranno a fondo perduto. L'Italia è stata l'unico Paese che ha richiesto l'intera quota del *recovery and resilience facility* (750 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione).

ha un rapporto tra dipendenti pubblici e cittadini estremamente basso rispetto alla media dei Paesi dell'Unione e purtroppo questo comporta difficoltà, anche per l'elevata età media dei l'elevata età media dei dipendenti statali e la loro scarsa formazione in progettualità. L'età media si aggira, infatti, intorno ai 50,7 anni e questo già fa capire che c'è una grande difficoltà nella capacità di formarsi per progettare e quindi per adeguarsi alle visioni degli investimenti che l'Europa fa per lo sviluppo dei vari Paesi. Inoltre, i tagli sono intervenuti in tutti i settori della pubblica amministrazione,

che se il Piano non dovesse essere approvato, ma dovesse essere restituito con delle osservazioni, la prima *tranche* dell'importo complessivo arriverà solo dopo

purtroppo l'erogazione dei fondi verrà interrotta. Pertanto rischiamo di compromettere inutilmente e gravemente il futuro delle prossime generazioni,

somma (i 191 miliardi) e che ci si ridimensioni sulla somma dei 68 miliardi che possono essere erogati a fondo perduto, privilegiando soprattutto le infrastrutture e l'intermodalità del Sud Italia che sono quelle che, purtroppo, possono veramente rilanciare lo sviluppo del Paese.

una sfida straordinaria da cogliere. Certo, una sfida ambiziosa - ce lo dobbiamo dire - sicuramente non semplice, men che meno scontata. Voglio partire da una considerazione: oggi l'Istat certifica che il livello di benessere nel nostro Paese è distribuito sempre meno equamente. In questa pandemia ci siamo entrati con forti disuguaglianze tra i livelli di inclusione e quelli di esclusione, l'abbiamo poi attraversata con differenze pesanti tra chi è stato più garantito e chi meno; ne usciamo sicuramente con quei divari che si sono allargati e approfonditi. Lo abbiamo detto, allora, più volte: non è più soltanto una questione di giustizia sociale; si tratta di precondizioni necessarie per noi per immaginare crescita e sviluppo del nostro Paese. Non c'è ripartenza senza recuperare i divari che oggi impediscono un accesso equo al Servizio sanitario nazionale, ai troppi giovani di laurearsi nei tempi e poi essere assorbiti nel tessuto produttivo, al Sud, ma non solo. E poi le donne, giovani e meno giovani, che, come abbiamo detto tante volte fino davvero a stancarci - sono la vera risorsa, anche dal punto di vista della crescita, rimasta oggi poco valorizzata e riconosciuta. Per questo è senz'altro un bene che donne, giovani e Sud siano stati scelti come i tre assi trasversali del Piano. Non siano adesso, però, il modo per disperdere queste risorse, proprio perché, al contrario, invece ne devono rappresentare quell'approccio multidimensionale che di questo piano rappresenta, appunto, il valore aggiunto. È fondamentale soprattutto in quelle aree - penso al Mezzogiorno, alle aree interne - dove, insomma, c'è più bisogno di coesione sociale e sostenibilità, dove va rafforzata l'offerta e la qualità di tutte le infrastrutture sociali, a cominciare ovviamente degli asili nido, ma non solo quelli, che rappresenta un investimento per l'occupazione femminile, certo, ma anche per il percorso scolastico dei nostri stessi bambini. Oggi la forbice del divario di genere sul mercato del lavoro continua ad allargarsi. Le cause sono le più diverse. Prime tra queste, quelle settoriali, quelle proprio legate alla pandemia perché servizi privati come commercio e turismo sono servizi a composizione prevalentemente femminile. E, allora, qui nessuna esitazione; lo ha detto il piano Colao, noi lo ribadiamo: bisogna investire pesantemente in quei settori a elevata presenza femminile, che tra l'altro saranno i primi a ripartire sicuramente, una volta terminata la pandemia. Ma non c'è solo questo. Molte donne hanno lasciato il lavoro perché i modelli sociali di riferimento ancora non consentono compatibilità tra vita privata e lavoro. Questo non è un effetto solo della pandemia. Se oggi si sacrifica il posto di lavoro pur di far fronte alle chiusure di scuole, servizi educativi, servizio a domicilio, il problema non è solo delle donne; è anche degli uomini, e sta nell'assenza di una condivisione degli oneri di cura tra uomo e donna, nel fatto che i percorsi di carriera delle donne sono più discontinui, precari e vulnerabili. Per far fronte a questo non bastano gli incentivi, men che meno se a pioggia. Serve una legge importante sulla parità salariale; serve soprattutto un piano per l'occupazione femminile di lunga durata e qualificata; serve un investimento senza precedenti in infrastrutture sociali, ma serve ancora e più di tutto - lo ribadiamo - la valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle politiche adottate. Per questo è necessario un osservatorio destinato allo scopo. O rompiamo questa spirale perversa oppure tutta l'Italia si ritroverà più debole sul lato dei diritti e ancora più povera sul lato della crescita; le due cose per noi non possono essere disgiunte. L'aumento dell'occupazione femminile - ricordiamolo sempre - avrebbe benefici enormi sul PIL, ma ne avrebbe anche per noi soprattutto sull'autonomia sociale e relazionale di tutte quelle donne che, anche per questo, oggi sono esposte a molestie, maltrattamenti, violenza in casa e sul luogo di lavoro. Autonomia e libertà sono gli unici, veri, efficaci antidoti alla violenza, ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ma se il *recovery plan* è un'occasione unica, oltre ai soldi servono le riforme, quelle strutturali, insieme alla capacità di gestire progetti nella fase esecutiva ma anche in quella di regolazione. Siamo nel mezzo di due trasformazioni che la pandemia ha accelerato e che qui mi limito ad accennare: transizione ecologica e digitale. Entrambe stanno cambiando modelli sociali di condivisioni e di lavoro, nonché sistemi di produzione e protezione. Non illudiamoci che basti evocare il cambiamento per vederlo realizzato o per vedere superato un modello di sviluppo che oggettivamente ha mostrato tutti i suoi limiti. La sostenibilità è centrale, ma questo non significa che sia destinata ad affermarsi. Non è affatto scontato che le trasformazioni siano di per sé eque, inclusive e democratiche. Per questo, soprattutto sul lavoro e sul *welfare* servono in questo momento una visione e una strategia per il futuro che non si limitino ai prossimi anni (quelli fino al 2026, per intenderci), ma progettino i prossimi decenni su sanità territoriale, scuole e servizi. La ferita aperta dal Covid è davvero la più profonda. Dunque, ripartiamo da *welfare* universalistico e diritto alla formazione costante e di qualità. Serve poi un ampio investimento sulle capacità dei lavoratori, non tornando indietro sulle misure di sostegno alla povertà, ma riformando ammortizzatori sociali e innovando gli strumenti e le politiche attive. Si è parlato poco - o meno del dovuto - delle risorse destinate alle periferie, alla rigenerazione urbana e all'*housing* sociale. Si tratta di un altro settore in cui transizione ecologica e inclusione si intrecciano, ma per farlo adeguatamente è necessario che le risorse si compattino e rispondano a un'unica regia. Infine, riprendo una cosa che ha ricordato il ministro Franco. Il Piano è uno strumento straordinario che deve funzionare accanto agli strumenti ordinari già previsti, tra cui fondi strutturali e fondi di coesione. Va invece assolutamente evitato che la spesa aggiuntiva per gli investimenti del Piano sia compensata al ribasso da una minore spesa ordinaria - questo è fondamentale - o che si traduca in infrastrutture sociali che poi non sono supportate da un investimento duraturo nel tempo, anche nel bilancio dello Stato. Mi sia consentita un'ultima considerazione sul ruolo della pubblica amministrazione. Va garantita una gestione adeguata dei progetti e per questo serve un coinvolgimento efficiente delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, e di personale formato e competente. Se questo si deve tradurre in un piano di assunzione anche al Sud, come è stato annunciato, passare da una puntuale verifica dei fabbisogni e da un aggiornamento delle dotazioni organiche degli enti a cui le nuove professionalità saranno destinate. L'Italia ha su di sé una grande responsabilità. Oggi che la posta in gioco è così alta abbiamo l'occasione di uscire dalla tentazione di incolpare l'Europa per qualsiasi cosa non vada nel nostro Paese, invece di entrare nel merito delle opzioni per il nostro futuro. Per questo abbiamo bisogno che soprattutto le forze politiche si mostrino capaci di leggere questo nostro tempo, rinnovando idee e priorità su cui investire. Il Partito Democratico non mancherà di far sentire le proprie proposte e la volontà di far sentire forte il suo contributo.

sia chiaro che oggi diamo il via a un Piano da circa 200 miliardi di euro che deve servire al rilancio dell'Italia intera, da Nord a Sud.

attenzione perché il *recovery fund* potrebbe anche diventare un gigantesco spreco e risultare del tutto inutile se dopo la spinta iniziale generata da questi fondi non seguirà un deciso cambio di rotta rispetto all'attuale immobilismo in cui versa la nostra Nazione. In un solo anno abbiamo operato scostamenti di bilancio per circa 180 miliardi di euro per fronteggiare la pandemia. Abbiamo dovuto farlo, è vero, ma è altrettanto vero che diverse di quelle risorse sono state sprecate dal presidente Conte perché è mancata una progettualità. Cosa è rimasto, infatti, di questo immane sforzo chiesto agli italiani? Qualche migliaia di banchi a rotelle e poco altro. All'Italia serve invece un cambio di mentalità e abbiamo una nuova possibilità che non deve essere sprecata. Il *recovery fund* ha regole rigide. I paletti dell'immediata cantierabilità dei progetti e il limite temporale dei lavori che devono essere terminati in cinque anni hanno permesso di inserire nel Piano solamente opere che sono effettivamente e immediatamente utili. La spinta al completamento dei corridoi TEN-T rientra in quest'ottica, così come il potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità, il dragaggio dei porti, gli investimenti per la messa in sicurezza delle principali infrastrutture idriche e la manutenzione delle strade provinciali della Penisola, specialmente nelle zone interne. Stiamo quindi probabilmente per uscire da un periodo buio e dobbiamo pensare al rilancio del Paese. Siamo uno Stato a forte vocazione turistica e per questo motivo occorre lavorare sulle infrastrutture perché dobbiamo soddisfare una clientela che è sempre più esigente. In quest'ottica abbiamo quindi indicato la necessità di allocare risorse per il sostegno e il rilancio del settore aeroportuale, in modo da garantirne la competitività a livello internazionale: porti, aeroporti e l'intermodalità per accedervi sono fondamentali per tutto il sistema Italia. Dobbiamo quindi darci un nuovo metodo di lavoro: l'azione deve essere incentrata sulle finalità corrette e sulla modalità di raggiungimento di queste che abbiano uno scopo e che siano sensate e prive di ideologie preconcette. Bisogna essere pratici per ottenere l'obiettivo in tempi rapidi: concreti, insomma. insomma. L'Europa finanzia opere che devono essere determinate in cinque anni: saranno marziani questi che l'hanno deciso, oppure dobbiamo chiederci noi perché in Italia, per terminare un esproprio, servano dai due ai dieci anni?

No, non è normale, non è normale per niente. E non fingiamo di non sapere a che cosa è dovuta la gran parte di questi ingranaggi così ingessati: è dovuta al codice degli appalti. Ecco quindi che occorre riformarlo ed è arrivato il momento di farlo non perché lo dico io, perché lo dice Campari; dobbiamo farlo perché sarebbe stupido semplicemente non farlo. Dobbiamo dedurre gli oneri burocratici e semplificare le procedure. Vogliamo ricordarci che abbiamo ideato il modello Genova, che siamo ci siamo liberati della burocrazia ed abbiamo ritrovato il lavoro e l'efficienza? Io credo semplicemente che dobbiamo svegliarci. Allo stesso modo, occorre liberarsi da quelle ideologie che rischiano di portarci dentro vicoli ciechi e di provocare effetti del tutto contrari a quelli che vorremmo invece avere. Faccio due esempi

Ma come pensiamo di rinnovarlo se diamo incentivi solamente per i veicoli ibridi ed elettrici? Quando capiremo che dobbiamo incentivare l'acquisto di veicoli di nuova costruzione, non inquinanti ovviamente, indipendentemente dal tipo di propulsione? seconda considerazione riguarda le autostrade. È stato detto che le nuove autostrade generano maggiore traffico inquinante. Ma se la costruzione di un'autostrada di 60 chilometri sostituisce un percorso di 125 chilometri inquineremmo di più o di meno secondo voi? Lo dico perché questo è il caso reale, esistente della Tirreno-Brennero, e se qualcuno mai non lo sapesse, adesso lo sa. Dobbiamo insomma affrontare il futuro in modo pragmatico. Il metodo Il metodo che stiamo importando dovrà servire da qui in avanti, anche per l'utilizzo dei fondi ordinari dello Stato. Si sono liberati capitali che erano stati impegnati a copertura di alcune opere finanziate con il *recovery e abbiamo chiesto che questi capitali siano reimpiegati per il finanziamento di nuove opere che non sono comprese nel Piano in esame. Dopo questa terribile crisi, dovremo far ripartire il mondo del lavoro anche con nuove opere pubbliche, andando a finanziare le grandi strade e le infrastrutture. Saremo protagonisti e responsabili nella gestione dei nostri fondi. Dobbiamo essere un esempio per l'Europa. La Lega ha l'ambizione di cambiare in meglio l'Unione europea ed è positivo aver sentito che il nostro Presidente del Consiglio mette finalmente l'Italia e gli italiani al centro della nostra azione politica. Con orgoglio e a testa alta. Signor Presidente, è passato ormai più di un anno da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia e da quando il Covid-19 è entrato prepotentemente nelle nostre vite, stravolgendo tutte quelle regole, quelle azioni, quei gesti quotidiani, quelle abitudini e quella serenità che oggi ci sembrano soltanto un lontano ricordo. Il Covid ha messo in ginocchio l'economia mondiale e l'Italia in Europa è stata la prima a dover fronteggiare tutte le drammatiche conseguenze che il virus si trascina dietro. Fu proprio allora, nella scorsa primavera, che il presidente Conte propose all'Europa un rivoluzionario concetto dello strumento di aiuto sotto forma di debito condiviso, impensabile fino a quel momento per un'Unione europea più vicina alla finanza che ai cittadini: il *recovery fund,* di cui oggi ci troviamo a discutere entrando nel merito delle schede proposte dal precedente Governo. *(Applausi)*. Dall'inizio della pandemia in quest'Aula abbiamo votato sei scostamenti di bilancio, per un totale di 165 milioni di euro; abbiamo altresì convertito diversi decreti-legge, tutti volti a supportare

ha l'occasione non solo di uscire dalla crisi, ma di riprendersi e competere per i primi posti tra i Paesi più importanti del mondo. Non solo. L'Italia ha la possibilità di mostrare al mondo che essa è capace di affrontare ogni tipologia di crisi futura, restando integra e pronta a reagire: un Paese resiliente. Come esponente del MoVimento 5 Stelle non posso che essere soddisfatta dei tre assi strategici che caratterizzano questa proposta: digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale sono sempre stati i pilastri dell'idea che abbiamo avuto per lo sviluppo del nostro Paese. Ho avuto il piacere e l'onore di essere la relatrice per la parte di questo Piano che riguarda l'8a Commissione, la Commissione lavori pubblici, e ritengo che la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che garantirà un notevole snellimento della burocrazia, l'innovazione del sistema produttivo, l'uso di energie da fonti rinnovabili per i trasporti e l'industria e la mobilità sostenibile, temi cardine del Piano, siano interventi che faranno da volano per il rilancio post pandemico del Paese. La riduzione degli oneri burocratici, la semplificazione delle procedure degli appalti, la riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, l'introduzione di meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma RFI e ANAS, la semplificazione delle procedure che rafforzano meccanismi di vigilanza meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti sono misure che certamente porteranno grandi risultati, proseguendo di fatto il lavoro già avviato dai decreti sblocca cantieri e semplificazioni. Non è pensabile, Presidente, parlare di ripresa e resilienza avendo un Paese che corre a due velocità due velocità diverse. Il Mezzogiorno corre a una velocità diversa rispetto al Nord Italia, così come le aree interne rispetto alla costa. Parlo di infrastrutture carenti, vetuste e incomplete, che limitano quel grande potenziale raggiungibile invece da un'Italia compatta. compatta. Nella relazione illustrata oggi troviamo il potenziamento degli snodi principali dell'alta velocità e dei territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne, e il rafforzamento del trasporto via mare per le isole, garantendo il regime di continuità territoriale. Una penisola come l'Italia, che da sempre è porto naturale dell'Europa, necessita di valorizzare i propri porti, specie quelli del Mezzogiorno, rafforzando le capacità di intercettare i traffici intercontinentali delle merci, e di un piano efficiente di sistema intermodale capace di smistarle lungo tutto lo stivale. Anche questo ovviamente la Commissione ha raccomandato al Governo. La sostenibilità ambientale, Presidente, è il cardine di tutta la programmazione, perché in un mondo ecologicamente insostenibile è la sopravvivenza dello stesso genere umano a essere messa in discussione. Senza transizione ecologica non ci sono altre transizioni che tengano; noi siamo l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo. Anche se non ce ne accorgiamo, noi siamo natura e, senza un ambiente sano, non ci sono né salute, né benessere, né tantomeno vita. Fuori da quest'Aula ci sono le nuove generazioni che da tempo protestano perché gli è stato rubato il futuro e a noi tocca provare a restituirglielo. Oggi assistiamo alla svolta verde di un intero continente e tutto il mondo è concentrato sui temi ecologici. I fondi che l'Unione europea ha voluto dedicare alla transizione ecologica sono il segno di quanto debba essere centrale questo aspetto. Senza mobilità sostenibile e senza efficientamento energetico degli edifici le nostre città continueranno a essere inquinate e gli italiani continueranno ad ammalarsi e a morire, anche oltre il Covid. Siamo un Paese con un patrimonio immobiliare di notevole spessore estetico e anche qualitativo, ma altrettanto "attempato" e non certo pensato per ottimizzare i consumi energetici. Lo stesso presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 22 febbraio scorso, durante la settimana parlamentare europea, ha sostenuto che un uso corretto dei soldi del *recovery fund* è quello di impegnarli nella creazione di nuovi posti di lavoro, gli stessi posti di lavoro persi durante la pandemia, e ha fatto un chiaro riferimento al settore edilizio, in relazione alla vetustà del patrimonio residenziale privato. Molti come me, in quell'istante, quando ascoltavano quell'intervento, hanno pensato al provvedimento superbonus 110 per cento e alla necessità di prorogarne la scadenza almeno al 2023, per garantire rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e quant'altro. *(Applausi)*. È notizia di oggi che il superbonus ha superato il primo miliardo di euro di lavori eseguiti ed asseverati. L'Italia e gli italiani hanno sempre dimostrato di saper reagire ad ogni crisi e calamità subita. La stessa cosa stanno facendo ora. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo resiliente e a tutti loro va espresso il nostro massimo rispetto. Questo documento è la via di accesso ad un finanziamento che non ha eguali nella storia del Paese e di certo aiuterà a trascinarci fuori dalla crisi, ma l'occasione unica che questa volta abbiamo è quella di fare riforme storiche, che il Paese aspetta da un trentennio. Allora, signor Presidente, che questo Piano nazionale sia davvero uno strumento di riforma, costellato

le due misure più importanti di questo Piano sono la transizione ecologica e la transizione digitale, soprattutto perché, se pensiamo alla quantità di risorse che drenano, il 57 per cento, ci rendiamo immediatamente conto dell'importanza dei due verticali, che peraltro, permeando tutti i settori dell'economia reale, possono essere ritrovati anche nelle altre quattro misure.

che qualificano questa strategia: il capitale umano e la sua manutenzione costante. Come ho detto più volte, i giovani potranno cambiare anche dieci volte mestiere. Pensiamo ai nuovi mestieri, che dovranno

tutti coloro che hanno perso il lavoro (mi riferisco agli ammortizzatori sociali e alla cassa integrazione) ma che sarebbe ora anche di accompagnare, con politiche attive, a nuovi mestieri.

italiano. Oggi, proprio per la dimensione piccola, che una volta era considerata un limite e un difetto, soprattutto nel processo di internazionalizzazione, essa rappresenta qualcosa di importante e e di unico, perché è molto più flessibile, molto più duttile e molto più pronta ai cambiamenti, chiaramente se aiutata da questa infrastruttura digitale. amministrazione che va verso i cittadini e non i cittadini che vanno verso la pubblica amministrazione. Qui c'è una vera e propria rivoluzione da affrontare. Io credo che ognuno di noi sia fortemente preoccupato su questo fronte, perché sburocratizzare, prima ancora di introdurre il digitale, è fondamentale e necessario per evitare una bomba digitale. Ho già utilizzato proprio questi termini più volte nei miei interventi. Una breve riflessione letteralmente piegato. Turismo e industria creativa italiana possono rappresentare il meglio del *made in Italy*, un termine del quale tutti noi ci riempiamo la bocca. Anche in questo PNRR è presente. Finalmente, con questa infrastruttura digitale, noi possiamo internazionalizzare quella piccola e media impresa. Possiamo credere fortemente in una crescita del PIL, rispetto all'ultimo dato del 2019, molto facilmente in un medio periodo periodo (neanche troppo lungo, perché il digitale dà risultati velocemente), di 3-4 punti di PIL: non è poco, sono quasi 50 miliardi

per settori produttivi: bisogna verticalizzarla per settori produttivi, che siano affiancati da *hub* digitali, con incubatori-acceleratori che servano ad indirizzare la finanza verso le attività più innovative, più meritevoli di essere accelerate verso il mercato. Insomma, un nuovo modello di economia che ibridi il privato e il pubblico. Mi rendo conto che non è semplice da scrivere, in un ginepraio di regole contrattuali, di logiche autorizzative e di rigidità burocratiche, ma è d'obbligo, perché abbiamo visto che le grandi imprese, quelle che Galbraith definiva le tecnostrutture, sempre più evolute, sovrastano le capacità delle burocrazie pubbliche e, in qualche caso, perfino dei Governi. Il risultato è che sempre più spesso i grandi gruppi si trovano ad affrontare temi che hanno risvolti pubblici, ma lo fanno senza argini. Pensiamo a tutto il mondo dell'economia privata, allo sfruttamento dei dati, il vero petrolio di questa economia, e ai risvolti del demanio pubblico digitale e, dunque,

ha detto che bisogna collaborare ad una sovranità tecnologica europea con la Francia e la Germania. Peccato che la Francia e la Germania abbiano già individuato le loro sedi per le agenzie nazionali dell'intelligenza artificiale in mentre l'Italia non l'ha ancora fatto. Non va dimenticato il piano delle relazioni internazionali che, nella fase della globalizzazione matura, contano sempre di più. Da qui derivano le ultime due considerazioni, che sono due nervi scoperti.

Grazie, la scienza e la tecnologia, che entrano prepotentemente nella politica e che richiedono sempre più competenze. Queste competenze inevitabilmente spostano tutto verso le cosiddette *élite* politiche. Qual è lo scoglio da superare? È quello di evitare il da superare? È quello di evitare il distacco del popolo dalla politica e, quindi, l'emergere del populismo, dando autorevolezza alla politica, attraverso la capacità di comprendere i contenuti tecnici e scientifici che, in queste due transizioni fondamentali del XXI secolo, richiedono prepotentemente competenze e professionalità.

per l'Italia, nel pieno di una crisi così dura, che mette impietosamente a nudo gli errori fatti in passato, dovuti all'egoismo e al cinismo di politiche sbagliate. Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare e di costruire un tempo nuovo, di rilanciare le nostre democrazie e i nostri ideali, di dare futuro e protagonismo alle nuove generazioni, che sono le più colpite e che hanno perso fiducia. La pandemia non ha solo allargato le diseguaglianze e le disparità che c'erano prima e che conoscevamo, ma ne ha create di nuove, scompaginando e aumentando le linee di frattura sociale. C'è un mondo che vuole esserci, che vuole avere voce, c'è una società da ricostruire per farlo, serve una visione, un'idea di società, non bastano misure tampone o emergenziali. C'è una grande domanda di cambiamento e noi dobbiamo esserne all'altezza. C'è una domanda di protagonismo di troppi che oggi sono esclusi da divari e sistemi chiusi e inaccessibili. Serve una nuova stagione di diritti e di riconoscimento. Ci sono oggi troppi lavoratori invisibili; penso agli autonomi agli intermittenti. Non basta dare un po' di sussidi e un po' di assistenza; servono diritti per costruire sviluppo. sappiamo - porta con sé non solo la crisi economica e la crisi sociale, ma anche una drammatica crisi educativa in un Paese come il nostro dove l'ascensore sociale è bloccato perché da troppo tempo il nostro sistema di formazione non è finanziato come dovrebbe essere. Eppure nel mondo i grandi Paesi sono quelli che investono in misura maggiore in istruzione pubblica e in innovazione. Eppure, nel tempo della continua rivoluzione tecnologica, sempre più per avere un lavoro serve competenza; il diritto alla competenza e il diritto al lavoro sono strettamente connessi. ragione dobbiamo rilanciare il diritto allo studio come motore di un nuovo modello di sviluppo perché ancora oggi è il più formidabile strumento di emancipazione in un Paese come il nostro, dove c'è un tasso insopportabile di abbandono e di dispersione scolastica, che colpisce soprattutto i bambini più svantaggiati, dove è troppo basso il numero degli immatricolati all'università, dei laureati e dei ricercatori, dove a laurearsi sono nella quasi totalità i figli di coloro che già sono laureati, dove per un ragazzo che viene da un istituto tecnico o professionale è difficilissimo accedere all'università. Sono muri che dobbiamo buttare giù e per farlo serve aumentare il numero delle borse di studio, allargare la *no tax area*, rafforzare il *welfare* studentesco. In un Paese come il nostro - dove chi insegna a scuola o fa ricerca in università o negli enti è mortificato da un precariato insostenibile che è nemico della qualità dell'insegnamento e della qualità della ricerca, dei bisogni degli studenti, della loro domanda di futuro e di protagonismo investire in istruzione, università e ricerca pubblica, non è una battaglia di settore o di categoria, ma una grande sfida per il ruolo del nostro Paese nel mondo, per il nostro futuro. Per tali motivi dobbiamo provare a legare i piani di ricostruzione, di cui oggi discutiamo, con delle riforme strutturali per rilanciare la scuola dell'inclusione: più classi con meno studenti, più spazi, più tempo scuola, più plessi anche nell'entroterra e nei quartieri difficili, dove la mancanza di finanziamenti li ha tolti, una nuova didattica, più insegnanti, più ore di sostegno, più attenzione ai bisogni educativi speciali dei ragazzi più fragili. Per questo serve una riforma del reclutamento nella scuola, nelle università e negli enti perché insegnanti e ricercatori sono una grande potenza civile che è indispensabile al nostro Paese *(Applausi)* e sconfiggere il precariato, valorizzarli e dare loro il riconoscimento e il ruolo che oggi manca è fondamentale per il nostro Paese. Presidente, così come per l'istruzione, la rinascita del nostro Paese passerà dalla cultura che è infrastruttura sociale, grande bene pubblico, capace di coesione e competitività. Per farlo dobbiamo finalmente mettere al centro il lavoro, approvare uno statuto dei lavoratori della cultura, dello spettacolo e delle arti performative, che permetta loro di non stare più ai margini. Per farlo, per far emergere i nostri talenti, dovremmo avere norme che permettano alle imprese culturali e creative di non essere più in balia di un sistema troppo chiuso da posizioni dominanti. Presidente - e concludo - cultura, istruzione sport sono un formidabile moltiplicatore, non solo di economia, ma di legami sociali, questo soprattutto nelle realtà dov'è più difficile vivere e dove noi dobbiamo tornare a dare protagonismo ai nostri ragazzi, e rappresentano

che rappresenta l'idea dell'Europa della solidarietà. Quel Next generation EU che rappresenta un'idea d'Italia, quella della nostra Repubblica, in cui ogni ragazza e ogni ragazzo venga messo nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita.

Signor Presidente, inizierò con i ringraziamenti al Governo che ci ha assistito durante i lavori di Commissione e ai due relatori Presidenti che hanno tenuto insieme tutto

ripresa e resilienza che licenzieremo domani con le risoluzioni. successo quattordici mesi fa e come l'inizio dell'emergenza sanitaria abbia sconvolto completamente le nostre vite. Abbiamo dovuto abbassare per forza di cose il punto di osservazione; c'è stata la paura, la malattia, molte volte purtroppo la morte e comunque sono cambiate tutte le nostre abitudini. Sintetizzo, perché penso che quello che sto per dire renda molto l'idea. Pensate al turismo: turismo vuol dire lavoro, lavoro, economia, vuol dire tutta la filiera, la cultura, la socialità, lo sport, la natura, la salute, il cibo, l'eccellenza, la felicità e la dignità. Vuol dire la dignità del lavoro e la felicità delle persone che ne

Con questo Piano e queste risorse importanti cerchiamo di contrastare la crisi che è seguita alla pandemia. Due terzi di questi fondi saranno da restituire e chi li dovrà restituire? Soprattutto i giovani, che sono uno degli obiettivi trasversali. Io avrei preferito vedere come obiettivo del Piano la centralità dei giovani, perché saranno proprio loro a portare il fardello sulle spalle, più di noi che forse non abbiamo tutta questa prospettiva e soprattutto abbiamo già vissuto gran parte della nostra vita. Noi abbiamo cercato di migliorare anche le misure per i giovani nel documento che abbiamo preparato. Nelle varie Commissioni sono stati toccati punti fondamentali.

in generale e fare in modo innanzitutto che non ci sia dispersione scolastica, perché tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che lasciano la scuola

e non in modo miserevole, ma sì da poter essere loro stesse costruttrici del futuro del Paese. Molte cose sono state inserite nel Piano, ma penso che lo sviluppo dei progetti che verranno attuati

sentire una grande responsabilità verso le nuove generazioni, facendo tutti gli sforzi possibili per garantire un po' più di salute di salute e di sviluppo anche alla generazione dei loro nipoti - questo lo dobbiamo loro - anche andando incontro a cambiamenti di abitudini, mettendosi in gioco e imparando cose che non hanno mai fatto.

migliori e più formati e dobbiamo alzare il livello di tutti, perché solo così potremo avere una società più sana e un'economia

Gli organi di stampa hanno riportato doviziosamente che il Presidente del Consiglio comunale di Ciampino, un esponente della Lega poi autosospesosi, avrebbe picchiato autosospesosi, avrebbe picchiato la moglie di fronte ai figli che erano in DAD. I Carabinieri e l'autorità giudiziaria stanno facendo gli accertamenti del caso,

sulle donne è una tragedia, ma lo è ancora di più se il presunto colpevole è anche un esponente delle istituzioni. Soprattutto, non è bello

la presidente del Partito Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non dicano niente su questa vicenda. Inoltre, il Presidente del Consiglio comunale

Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che non bisognerebbe fare questi interventi, perché in situazioni dovremmo prestare un'attenzione particolare e le cose dovrebbero risolversi diversamente da come effettivamente stanno, scorso ho depositato un'interrogazione riguardante i gravi eventi sismici del 2016 - purtroppo parliamo ancora di terremoto - che hanno colpito il Centro Italia, interessando in questo caso anche il Comune di Tolentino (Macerata). Evidenzio l'importanza di questa situazione per chiedere lo snellimento delle procedure atte a consentire una sistemazione rapida e dignitosa ai terremotati, oggi ancora in attesa. Provo a ricostruire brevemente i fatti. L'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, stabilisce che le Regioni interessate dagli eventi sismici, invece di procedere alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (le famose SAE), avrebbero potuto acquisire abitazioni da assegnare in comodato d'uso gratuito ai residenti ai residenti che abbiano avuto edifici distrutti, danneggiati o dichiarati inagibili. Fin qui tutto bene. Il dipartimento della Protezione civile emesso l'ordinanza n. 510, destinando 20,85 milioni di euro a Tolentino per la realizzazione di nuovi immobili in sostituzione delle SAE. La consegna delle unità immobiliari era stata stimata al 31 agosto 2019, ma ad oggi rileviamo che sono stati consegnati solo 21 appartamenti su 45. Inoltre, questi ultimi non sono nemmeno completi delle dotazioni che erano previste.

bisognerebbe preoccuparsi di risolvere la situazione che fino a un certo punto era stata portata avanti correttamente. Avviandomi alle conclusioni, a mio avviso risulta necessario assumere immediatamente idonee iniziative affinché siano condotte indagini approfondite

vorrei evidenziare in Senato un caso emblematico di dissesto idrogeologico che ha raggiunto la ribalta nazionale e desta forti preoccupazioni: la riattivazione di una grande frana, situata sul versante sudorientale del Monte Saresano, nei pressi di Tavernola Bergamasca sul lago d'Iseo. Si tratta di una frana di scivolamento planare che interessa un versante con calcari marnosi stratificati a franapoggio, interessato da un fronte di cava non più attivo, incombente sulla strada litoranea del lago d'Iseo. Il volume mobilizzato è enorme, pari a circa due milioni di metri cubi. La frana è in progressivo rallentamento e adesso si muove a una velocità inferiore a un centimetro al giorno, dopo aver toccato punte di quasi quattro centimetri al giorno alla fine di febbraio. Sono stati valutati i possibili scenari. In quello peggiore, la frana si propagherebbe fino al lago d'Iseo, generando così un'onda anomala. che potrebbe potenzialmente raggiungere le aree limitrofe dell'abitato di Tavernola Bergamasca, la costa orientale del monte Isola, oltre ad altre località rivierasche. È tuttavia presumibile che un evento di tale portata sia preceduto da un'accelerazione dei movimenti rilevabili dal monitoraggio in atto, garantendo un sufficiente preavviso per le necessarie procedure di protezione civile. Purtroppo, il dissesto idrogeologico in Italia interessa il 91 per cento dei Comuni, con alluvioni quotidiane e 620.808 frane censite (i due terzi di tutte quelle europee). Le cause del dissesto idrogeologico sono molteplici: le condizioni geologiche, l'errato uso del suolo, il degrado del reticolo idrografico minore, il continuo consumo di suolo e, negli ultimi tempi, il cambiamento climatico. La causa principale è tuttavia di natura sociale e culturale: la scarsa attenzione dedicata al problema, la memoria corta sugli eventi disastrosi e l'insufficiente educazione in materia sono tutti fattori che hanno portato inevitabilmente a distorsioni nella pianificazione dello sviluppo del territorio. Il problema si risolve con una scaletta di priorità magica: conoscenza, pianificazione, gestione e manutenzione del territorio. Signor Presidente, mi riallaccio all'intervento fatto questa mattina dal collega Bagnai

per motivi ideologici, per questioni di opinioni. Questo colosso multinazionale, più potente di molte ditte manifatturiere, decide cosa si può vedere e cosa non si può vedere. La logica la quale questo sarebbe come un *club* privato, dove ciascuno decide chi può parlare e chi non può, non regge.

impongono, per l'appunto, la *par condicio* specialmente in periodi elettorali. Quindi, se si può imporre alle televisioni private, si può - e a questo punto si deve - imporre una disciplina di salvaguardia del libero dibattito anche a questi colossi del *web,* che tra l'altro, in pratica evadono le tasse nel nostro Paese, anche quando gli inserzionisti sono italiani, si rivolgono a un pubblico italiano e si allacciano a video italiani. italiani. Mi associo a quello che tanti hanno detto, da tante provenienze politiche, ideologiche e professionali diverse: bisogna che ci sia un'iniziativa - mi appello al Presidente del Senato, che so sensibile al riguardo, per aver sottolineato la gravità della cancellazione degli *account* di un senatore o forse più di uno - perché è davvero importantissimo che continui a essere garantita la libertà di espressione a tutti, quali che siano le loro opinioni. Grazie,

la scorsa settimana abbiamo celebrato la Giornata mondiale dell'acqua quale bene fondamentale per la vita dell'uomo, in quanto elemento che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze dagli sprechi e dall'inquinamento. Quando penso a questi temi non posso non collegarli al mio territorio, dal quale ho raccolto le ennesime preoccupazioni di molti cittadini residenti nel basso Piemonte e sugli appennini liguri. depositato la terza interrogazione sulla questione grandi opere, in particolare Terzo valico, una linea merci che dovrebbe collegare il porto di Genova con Tortona alla modica cifra di 6,8 miliardi di euro per 53 chilometri di rotaie e

tutto venisse svolto nel pieno rispetto delle regole ambientali e della tutela, della salute e sicurezza dei lavoratori. Quando si parla di grandi opere, si parla sempre di grandi benefici economici e lavorativi per i territori; a me, però, duole constatare che tutto ciò non sta avvenendo, anzi. Non stanno avvenendo né il rispetto dell'ambiente, né la difesa delle fonti appenniniche e delle falde acquifere. La scorsa estate interi paesi sono rimasti senza acqua potabile, i residenti tra i Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Rivalta Scrivia hanno visto visto le loro cantine allagate, a distanza di mesi dagli eventi alluvionali, perché in entrambi i casi pare che i lavori abbiano intercettato la falda, prosciugandola nel primo caso e ostruendola nel secondo. Non si stanno tutelando adeguatamente i lavori all'interno dei cantieri del Terzo valico; si contano infatti diversi morti e molti incidenti gravi, che hanno portato a mutilazioni e invalidità permanenti; l'ultimo si è verificato proprio venerdì scorso, quando un operaio schiacciato da un'escavatrice ha perso la gamba destra, e i medici stanno lottando per salvargli almeno l'arto sinistro da probabile amputazione. Per non parlare delle aziende dell'indotto che hanno aperto procedure di licenziamenti: quindi, si parla di lavoro per il territorio, però questo lavoro sta finendo. Non si stanno verificando i benefici economici per i territori coinvolti: nel 2018 siamo riusciti a far destinare due milioni di euro per la progettazione del nuovo parco smistamento merci di Alessandria, opera collegata sempre al Terzo valico, e qui chiedo come siano state destinate quelle somme o se nel frattempo siano state utilizzate, perché ad oggi non è dato sapere.